nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 14 ottobre. ottobre. Oggi pomeriggio, come già stabilito, il Ministro dell'istruzione renderà un'informativa sull'avvio dell'anno scolastico, cui seguiranno gli interventi dei Gruppi per circa 2 ore e 50 minuti. A conclusione del dibattito, su richiesta del Gruppo della Lega Nord, si svolgeranno interventi relativi all'assassinio a Novi di Modena di una donna di origine pakistana da parte dei familiari. Si passerà poi - ove possibile - all'esame del disegno di legge sul divieto di propaganda elettorale per persone sottoposte a misure di prevenzione. In apertura della seduta antimeridiana di domani, sarà data la parola a un rappresentante del Gruppo del Partito Democratico che ha chiesto di intervenire su alcune dichiarazioni rese giovedì scorso dal senatore Ciarrapico nel corso del dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Potranno seguire interventi da parte di altri Gruppi. Sempre nel corso della seduta antimeridiana di domani, che terminerà alle ore 12,30, oltre all'eventuale seguito del disegno di legge in materia di propaganda elettorale, sarà esaminato il disegno di legge recante modifiche al codice civile in materia di potestà genitoriale. La seduta antimeridiana di giovedì 7 ottobre e, se necessario, la seduta pomeridiana di domani potranno essere sconvocate in relazione all'andamento dei lavori

si svolgeranno l'informativa del sottosegretario Bertolaso sulla ricostruzione post-terremoto in Abruzzo e i successivi interventi dei Gruppi per 5 minuti ciascuno. È stata inoltre acquisita la disponibilità dello stesso Sottosegretario alla Protezione civile a rendere - presumibilmente nel pomeriggio di giovedì 21 ottobre - un'informativa all'Assemblea sulle conseguenze dell'alluvione di Messina dello scorso anno. Il Gruppo di Futuro e Libertà ha chiesto poi di poter discutere della questione dei rifiuti a Napoli, eventualmente anche in Commissione. Per quanto riguarda il calendario della prossima settimana, martedì 12 ottobre, alle ore 16, prima che abbia inizio la seduta pomeridiana, si svolgerà nell'Aula del Senato la commemorazione solenne del senatore a vita, presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga, alla presenza del Capo dello Stato e delle più alte cariche istituzionali. La cerimonia si articolerà nell'intervento della Presidenza e quindi dei rappresentanti dei Gruppi. Ciascun Gruppo avrà a disposizione 10 minuti, eventualmente divisibili in più interventi. Sempre martedì 12 ottobre, alle ore 18, sarà discussa la relazione della 14a Commissione permanente sui rapporti tra Commissione europea e Parlamenti nazionali. Si è proceduto alla ripartizione dei tempi del dibattito, che si concluderà entro la seduta stessa con la votazione di un documento. Nelle due sedute di mercoledì 13 ottobre sarà posto all'ordine del giorno il documento recante la Decisione di finanza pubblica. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi secondo un criterio non strettamente proporzionale, tenendo conto delle richieste di alcuni Gruppi di opposizione. In ogni caso, le dichiarazioni di voto e il voto finale avranno luogo nella seduta antimeridiana di giovedì 14 ottobre. Riprenderà quindi, nella stessa seduta, la discussione dei disegni di legge di riforma della professione forense. si procederà al rinnovo delle Commissioni permanenti nell'intervallo tra le due sedute di mercoledì 13, negli orari che saranno successivamente comunicati.

Illustre Presidente, onorevoli senatori, avviare un anno scolastico è sempre un'operazione di estrema complessità. Quest'anno, peraltro, la sfida era ancora più impegnativa. Si trattava, infatti, di applicare per la prima volta una riforma organica che cambia, anzi ha cambiato, completamente il volto della scuola superiore italiana. Nuovi indirizzi, nuovi orari, una riorganizzazione totale dell'offerta formativa attesa da decenni e poi, come ogni anno, i soliti adempimenti: gli uffici regionali erano chiamati ad occuparsi di rispondere alle domande di mobilità del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e poi gli organici, le cattedre, le immissioni in ruolo, le supplenze. Insomma, una mole di lavoro considerevole, che è stata svolta però in maniera esemplare. credo che la sfida di aprire regolarmente l'anno scolastico sia stata vinta. Non sono mancate certo, come sempre, polemiche e contestazioni, ma sono state nella sostanza smentite le pessimistiche e spesso strumentali previsioni di un caotico e magari ritardato inizio dell'anno scolastico per effetto dell'applicazione dell'articolo 64 della legge n. e degli interventi legati all'attuazione e alla messa a regime della riforma del primo e del secondo ciclo. Colgo dunque l'occasione per ringraziare da questa autorevole sede istituzionale le strutture ministeriali, gli uffici scolastici regionali e territoriali

soprattutto a questa maggioranza di uomini e donne, dirigenti scolastici, insegnanti motivati, vada rivolto il nostro ringraziamento quando si parla di scuola italiana. Ma prima di entrare nel merito delle misure che hanno accompagnato necessariamente l'entrata in vigore e poi l'attuazione della riforma della scuola superiore in quest'anno scolastico, non voglio eludere il tema delle risorse attorno al quale sono nate polemiche aspre, che hanno diviso e continuano a dividere gli schieramenti e anche il Paese. Voglio partire da un'analisi, credo oggettiva, contenuta all'interno di un documento di inquadramento del sistema scolastico: mi riferisco al Libro bianco redatto durante il precedente Governo dal quale risulta, da una lettura attenta, evidente a tutti una sproporzione nella gestione delle risorse tra l'impiego del 97 per cento delle medesime per le spese correnti ed il risultato di riservare un misero 3 per cento alla qualità, agli investimenti. Si è molto discusso sull'entità dei tagli al personale docente e amministrativo. Si è più volte lamentata una cura eccessiva, una razionalizzazione non sopportabile per la scuola. Nulla di tutto ciò, perché, se si va a vedere effettivamente la portata di quella manovra, si scopre che a fronte dei 42.000 tagli previsti dal precedente anno, ben 32.000 erano

di una manovra che continuo a pensare assolutamente sopportabile e indispensabile per invertire un *trend* di crescita della pianta organica non proporzionato al fabbisogno effettivo di di posti da insegnante o da dirigente scolastico richiesti dalla scuola italiana. Voglio ricordare

e non più alle spese fisse. I primi risparmi racimolati hanno consentito agli insegnanti di non perdere gli scatti di anzianità:

170 nuovi posti di dirigente scolastico, ed è stato inoltre bandito un concorso per dirigente scolastico (per la prima volta sulla base di prove selettive e non più soltanto con concorso per titoli) per 2.800 posti.

constatare quanto vi sto dicendo, ovvero che sono stati immessi in ruolo 3.500 nuovi insegnanti di sostegno in più rispetto all'anno precedente. Credo che anche questo sia un segno importante da sottolineare. Ciò non significa aver risolto tutti i problemi o negare

distribuiti posti di lavoro che nei fatti si sono tradotti in posti di attesa nelle graduatorie. Cercare di ribaltare la realtà, attribuendo ad un provvedimento dell'attuale

dell'opposizione. E allora io invito ad analizzare, a riflettere, a dibattere su un tema delicato come quello della scuola (che appartiene al Paese e non è né di destra né di sinistra) non con la lente dell'ideologia o del pregiudizio, ma andando a guardare i numeri. Lì si scoprirà che ci sono sicuramente delle ombre, ma anche molte luci. Mi riferisco ad alcuni provvedimenti

Veneto, Lazio), con ciascuna delle quali sono stati siglati accordi per 7, 10 o 20 milioni di euro, a seconda dei casi, e si è sicuramente cercato - e in parte ci siamo riusciti - di alleggerire la situazione dei precari. È chiaro che tale situazione non è stata risolta; è chiaro che il fenomeno del precariato resta sullo sfondo e resta un problema enorme per la realizzazione dei giovani, per la loro autonomia decisionale, per la loro prospettiva di crescita, di carriera e di autonomia dalla famiglia. Ma questo non è - lo ribadisco - il frutto di una cattiva finanziaria, bensì bensì è imputabile, credo, ad un sistema che, per troppi anni, non ha calcolato i fabbisogni di posti di lavoro (quindi di insegnanti) della scuola. Questo ha determinato da parte delle università,

Questo Governo ha voluto innanzitutto non essere corresponsabile dell'insorgenza di nuovo precariato. Per questo abbiamo cominciato a governare i numeri e a cambiare il regolamento sulla formazione iniziale dei docenti. iniziale dei docenti. Sappiamo che non può esistere una buona scuola senza dei bravi insegnanti: se è vero che le idee camminano sulle gambe degli uomini, la scuola cammina sulle gambe degli insegnanti. Rafforzare queste gambe è stato allora il primo obiettivo che ci siamo posti, con un nuovo regolamento per la formazione iniziale che prestasse attenzione alla qualità della didattica e alla qualità dell'insegnante: non solo sapere e conoscere la singola materia, ma anche saperla insegnare. In che modo? Attraverso il tirocinio: da uno studio teorico e, dall'altro, attraverso molte ore di lezione e di pratica nelle classi, con un docente *tutor* destinato ad accompagnare il percorso formativo e la pratica del giovane insegnante. abbiamo rivolto attenzione alla disabilità. Abbiamo disegnato un nuovo tipo di docente, in grado di padroneggiare la propria disciplina, ma anche - ed è la prima volta in Italia - di avere una preparazione di base sulle disabilità. Noi non abbiamo formato solo gli insegnanti di sostegno, ma abbiamo preteso che tutti gli insegnanti avessero una particolare attenzione e una particolare preparazione di base sulle disabilità. Ci siamo preoccupati che i nuovi insegnanti

è evidente che non c'è una piena sintonia fra coloro che iniziano il percorso all'interno delle nuove facoltà di formazione degli insegnanti e coloro che poi si laureano,

Inoltre, se da un lato, abbiamo garantito gli scatti di anzianità, dall'altro pensiamo che un sistema di formazione veramente qualitativo debba

per individuare una via che possa essere il più possibile condivisa: si può trattare di una strada contrattuale o normativa, ma certamente dobbiamo pensare alla valorizzazione del corpo insegnante.

formata da 20 alunni! Ebbene, ho cercato di capire se questa rappresentazione corrispondesse al vero oppure fosse - come ritenevo - un po' ingigantita. Ancora una volta vengono in aiuto i numeri. Per quanto riguarda le classi sovraffollate, si tratta di un problema reale, ma di dimensioni molto più modeste di come taluni lo dipingono. Le classi costituite da un numero di alunni superiore a 30 (si fa presente che esse sono esclusivamente quelle dell'istruzione secondaria superiore) rispetto al totale delle classi rappresentano lo 0,4

con più di 20-25 alunni; tuttavia credo abbiano fatto bene il Governo e, soprattutto, la Conferenza Stato-Regioni a trovare un accordo sul dimensionamento scolastico. in molti casi forse è meglio avere una classe sovraffollata piuttosto che tenere in funzione una scuola pericolosa, non sicura. Quindi, il dimensionamento scolastico, che tra l'altro (come sottolineato dalla Conferenza Stato-Regioni) è di competenza degli enti locali, è un atto dovuto e doveroso se vogliamo garantire un'edilizia scolastica conforme alla normativa europea, nella quale non vi siano rischi, non solo con riferimento agli elementi strutturali, ma anche agli elementi non strutturali. Purtroppo il nostro Paese è distante dal raggiungimento di questo obiettivo. Sottolineo poi che per il Governo l'edilizia scolastica per il Governo l'edilizia scolastica costituisce una priorità nazionale, tanto che fin dall'avvio della legislatura ci siamo attivati con numerose iniziative, anche di sostegno finanziario, dirette a favorire i compiti degli enti locali. come dicevo, abbiamo attivato un tavolo tecnico con la Conferenza Stato-Regioni per la condivisione dell'anagrafe, perché vi era un problema di aggiornamento e di informatizzazione dell'anagrafe sull'edilizia scolastica vi era anche un problema legato al completamento dei dati. Avevamo a disposizione, infatti, solo i rischi relativi agli elementi strutturali dopo la vicenda dolorosissima di Rivoli, ci siamo accorti che l'anagrafe non conteneva i rischi riferiti agli elementi non strutturali. quindi proceduto con un lavoro sinergico con le Regioni, con gli uffici scolastici regionali e anche con i Comuni e le Province, a seconda della competenza sulla scuola primaria secondaria di primo e secondo livello, a fare anche dei sopralluoghi. Pertanto, l'80 per cento del patrimonio edilizio scolastico italiano è stato oggetto di sopralluogo con tecnici del Comune o della Provincia, a seconda dei casi, con un referente regionale e anche con un referente del Ministero delle infrastrutture e del Ministero della pubblica istruzione, al fine di avere al fine di avere una ricognizione puntuale della situazione prima di decidere dove andare ad investire. È chiaro che il fabbisogno è molto oneroso, nel frattempo è stato però attivato il piano straordinario di messa in sicurezza delle scuole nelle zone a rischio sismico. Si è disposto l'utilizzo di 20 milioni annui per la sicurezza delle scuole, derivanti dai risparmi sulle cosiddette spese per la politica. Si è proceduto alla definitiva assegnazione agli enti locali, attraverso un accordo con l'INAIL, di 70 milioni di euro; sono stati opportunamente reperiti un miliardo di euro dal fondo FAS per l'edilizia scolastica, di cui 226 milioni sono serviti alla ricostruzione delle scuole in Abruzzo e, del resto, dopo faticose trattative, è stato quantomeno ripartito il primo stralcio, di circa 300 milioni, stiamo procedendo al secondo stralcio, in accordo con il ministro Matteoli e con il sottosegretario Mantovani, al fine di posizionare queste risorse, dando la priorità agli interventi più urgenti, così come risulta dall'anagrafe ormai aggiornata. Come dicevo, oltre l'80 per cento degli edifici scolastici sono stati visitati da squadre tecniche appositamente costituite, che hanno verificato tutti gli elementi di pericolosità di carattere non strutturale. Con i primi risultati è stato predisposto un piano straordinario d'intervento. La Commissione bilancio della Camera sta peraltro procedendo alla ripartizione, a parte il miliardo di euro, di altri 300 milioni. È chiaro che non sono cifre esaustive e sufficienti per far fronte al fabbisogno di miglioramento dell'edilizia scolastica; sono però cifre importanti che, se verranno compartecipate dagli enti locali, potranno produrre un effetto moltiplicatore e diventare somme ancora più ingenti. La difficoltà sta nel velocizzare i tempi d'impiego di queste risorse, però credo che, anche in fase di stesura del piano per il Mezzogiorno - ne abbiamo già discusso con il ministro Tremonti e con il ministro Fitto liberare risorse per migliorare in modo particolare il patrimonio edilizio scolastico del Mezzogiorno, e stiamo trovando anche alcune

si tratta di orientare le proprie risorse dando la priorità assoluta a questo tipo di investimento. Si tratta anche in alcuni casi di decidere se sia più conveniente la ristrutturazione di una scuola fortemente fortemente disagiata e compromessa, o la costruzione di un nuovo polo scolastico; sicuramente l'investimento in questo settore è sacrosanto e assolutamente urgente.

parlare della scuola digitale, oggi presente solo marginalmente nelle nostre scuole, il 15 per cento degli alunni oggi può disporre della cosiddetta LIM, la lavagna interattiva multimediale: certamente stiamo svolgendo svolgendo azioni importanti in questa direzione, anche con l'aiuto del Ministero della funzione pubblica e di importanti aziende internazionali. Il piano di diffusione delle lavagne interattive multimediali infatti procede e, alla fine di quest'anno scolastico, saranno oltre 40.000 le classi dotate di una lavagna interattiva interattiva multimediale; un milione di studenti potrà apprendere le diverse materie attraverso questa nuova tecnologia e sono già stati formati 300.000 insegnanti per l'utilizzo di questo nuovo metodo. È evidente che ci troviamo in una fase di *start up,* cioè cioè ancora iniziale, ma comunque credo si tratti di un fatto importante, anche perché l'obiettivo è di far sì che la rivoluzione digitale tocchi anche le famiglie; sostanza, poter seguire l'andamento scolastico del proprio figlio attraverso Internet, consultare la pagella, prenotare colloqui con i professori, ricevere un sms quando il figlio è assente da scuola. Insomma, è destinato a finire anche uno dei rituali più longevi che si consuma ogni giorno nelle nostre scuole, l'appello, e attraverso la carta dello studente, che ogni alunno già da anni da anni possiede, si potrà entrare ed uscire da scuola ed essere registrati automaticamente. In questo caso, quasi la metà delle scuole superiori è stata dotata degli strumenti necessari. Quindi, si tratta di un percorso ancora lungo, che abbiamo appena avviato; un percorso che

e cercato di potenziare il sistema di valutazione. È noto che da tempo esiste l'INVALSI, un'agenzia di valutazione e di somministrazione dei test.

verificare precisamente l'andamento dell'apprendimento e della qualità dell'istruzione nelle scuole prese a campione.

l'istituzione di un'agenzia deputata alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti e attraverso sperimentazioni già messe in campo per comprendere qual è il meccanismo incentivante premiale migliore (se

In conclusione, mi sento di dire che il piano di razionalizzazione era già stato scritto nel Quaderno bianco. Ci siamo assunti la responsabilità di attuarlo.

peraltro convinta che si possa ridurre il tema della scuola esclusivamente ad una questione di risorse: è un problema di riforme, ed è legato alla modalità con stesse vengono spese. Se riusciamo ad evitare gli sprechi, a cambiare le regole, a migliorare l'impianto formativo per la scuola

a medio termine consegnerà al Paese sicuramente una scuola migliore.

Gelmini una domanda su una questione specifica, sulla quale mi auguro di poter avere una risposta precisa, esauriente e priva della genericità del suo ho chiesto di prendere la parola per chiederle notizie sui provvedimenti relativi alla riduzione dell'orario degli istituti tecnici, in relazione alla nota sentenza del Consiglio di Stato. però parlare tra breve, perché il suo intervento mi sollecita a fare anche delle considerazioni di carattere generale sull'apertura dell'anno scolastico e un po' sul bilancio di due anni e mezzo di governo del Ministero dell'istruzione. Vede, la settimana passata, il presidente Berlusconi è venuto in Senato, dopo essere stato alla Camera, per chiedere la fiducia sostanzialmente su cinque questioni che aveva già proposto

Governo; due anni e mezzo al termine dei quali non ha potuto portare alcun dato significativo di risultati su riforme, interventi, miglioramento complessivo della situazione del Paese.

a suoi interventi, e debbo riconoscere - e sul piano personale mi fa piacere dargliene atto - che lei espone sempre con estrema cortesia e con un tratto di grande signorilità una serie di di buone intenzioni, di buoni propositi ed anche di buoni sentimenti rispetto alla nostra scuola.

Lei sa bene che in una simile congiuntura politica tale rinvio, al quale ovviamente - altrimenti non sarebbe stato possibile - ha collaborato la sua maggioranza, significa sostanzialmente l'affossamento

un sostanziale nulla. ha dichiarato che la addolora sentir parlare di tagli) di migliaia di posti di lavoro di personale e di insegnanti. Anche questo anno scolastico 2010-2011 inizia sotto il segno della mancanza di risorse adeguate a garantire il funzionamento minimo degli istituti scolastici: mancanza di supplenti, riduzione degli orari, conseguente venir meno della continuità didattica e con la perdita di migliaia di posti di lavoro, che non diminuiscono ma addirittura aumentano il fenomeno del precariato. Il riordino del sistema scolastico, realizzato dal suo Ministero con vari regolamenti ministeriali, sostanzialmente è una mera riorganizzazione necessaria per adeguare il sistema scolastico ai tagli decisi dal Ministro dell'economia. Questa è la logica che sovrintende a tutta la regolamentazione del suo Ministero. Come noi possiamo parlare di riforma, se tutte le decisioni dipendono esclusivamente da precedenti decisioni di carattere finanziario che hanno impoverito strutturalmente la scuola? È vero, come lei ha detto poco fa,

A conferma di questa politica di disinvestimento, i recenti regolamenti di riordino degli istituti professionali (che è la questione che le ho sollevato all'inizio) prevedono una ridefinizione al ribasso in termini di strutture e di organici. Signora Ministro, questa è la questione specifica sulla quale le chiedo di esprimersi. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del suo Ministero, quindi un suo ricorso, avverso un'ordinanza del TAR, con il quale lei chiedeva la sospensione dei provvedimenti relativi alla riduzione delle risorse complessive. Il TAR aveva bocciato il provvedimento del Ministero, il Ministero aveva ricorso al Consiglio di Stato e il Consiglio ha bocciato la tesi del Ministero. Ora, davanti a una decisione del Consiglio di Stato

la decisione del Consiglio di Stato per il Ministero è assolutamente irrilevante e che la notizia che il Ministero debba rifare le misure organizzative contro le quali il Consiglio di Stato si è espresso è una decisione priva di ogni fondamento. qui abbiamo anche a che fare con principi generali di uno Stato di diritto. Esistono due decisioni dell'autorità giudiziaria amministrativa. La decisione del Consiglio di Stato, come lei sa, è definitiva. Ma per quale motivo il Ministero non deve dar seguito a una decisione precisa, con la quale il Governo viene dal Consiglio di Stato impegnato a prendere misure....

ma l'argomento, signora Ministro, come lei sa, è talmente serio e talmente consistente che avrebbe meritato uno sviluppo ben più lungo dei sette minuti preventivati. La prego soltanto di voler essere precisa su quelli che sono i motivi per i quali il Governo ha ritenuto di non dare esecuzione, prima alla decisione del TAR e poi alla decisione del Consiglio di Stato.

il suo intervento i cui contenuti, devo dire molto generici (spiace doverlo ribadire), confermano ancora una volta le nostre preoccupazioni e il nostro disagio.

sia con riferimento alla qualità dell'offerta formativa e alle condizioni in cui si opera, sia con riferimento ai livelli occupazionali. Tale situazione, com'è noto, sta generando forti tensioni e grande disorientamento nel mondo della scuola. Quella che oggi vuol farsi passare per una riforma, e che ci trova in quest'Aula impegnati a dibattere, è piuttosto un preciso disegno irresponsabile di smantellamento della scuola pubblica. L'inizio dell'anno scolastico, del resto, ha già anticipato gli effetti devastanti della vostra riforma, di questa riforma, che solo formalmente - non ci stancheremo mai di dirlo - porta il suo nome, trattandosi di una riforma connessa ad una manovra fortemente voluta dal ministro Tremonti; una riforma finalizzata ad assicurare solo risparmi al bilancio dello Stato e ad operare tagli indiscriminati e scellerati, senza alcuna considerazione nel merito per il progetto educativo - sì, il progetto educativo - e con conseguenze davvero devastanti se si pensa a tutti gli operatori della scuola e, soprattutto, agli studenti. Tutto questo ovviamente è in perfetta sintonia - ci teniamo a sottolinearlo - con l'azione politica complessiva dell'attuale Governo, se si fa riferimento anche ad altri interventi, come quello nel campo della cultura. In questo quadro, signora Ministro (è questa la nostra maggiore preoccupazione), la scuola rischia purtroppo, nel più breve tempo possibile, di essere inesorabilmente destinata a non riuscire più ad assolvere ai propri compiti istituzionali: faccio riferimento ovviamente a quelli della diffusione delle conoscenze e, soprattutto, a quelli della formazione e della crescita. Noi siamo convinti che dietro ogni riforma, signora Ministro, ci debba essere un'idea, un'idea vera;

Non le sfuggirà che tutta l'esperienza di collaborazione dei docenti, che via via ha trovato maturazione nel tempo pieno, è stata estesa a tutta la scuola, diventando patrimonio ineludibile dell'intera istituzione scolastica. Non le sfuggirà altresì, signora Ministro, che la pluralità del corpo docente ha permesso al corpo docente stesso di approfondire la conoscenza delle diverse discipline, rendendo l'intera istituzione scolastica una vera e propria comunità di conoscenza. Nonostante ciò, il Governo ha voluto invece solamente un ritorno al passato, che permettesse di ottenere nuovi risparmi ai danni della già tartassata scuola pubblica, cioè di fare cassa, per usare un'espressione più comune. Ma le sembra questo, signora Ministro, il modo migliore di approcciarsi a tematiche così delicate? Ma ha mai fatto un giro conoscitivo nelle scuole? Se almeno questo avesse fatto, forse, piuttosto che liquidare l'intera riforma in tal modo, si sarebbe accorta che la scuola ormai non ha più neanche i fondi per sopravvivere: altro che progetti educativi! Si è mai preoccupata in questi anni di garantire la qualità della scuola pubblica? Si è mai preoccupata di avere a cuore il progetto formativo scolastico? Si è mai preoccupata di lavorare per adeguare la scuola italiana agli standard europei? Per capire realmente di cosa ha bisogno la scuola, bisognerebbe entrarci dentro, viverla con i professori, farsi raccontare da loro le loro esperienze ed utilizzare la loro esperienza affinché il servizio dell'istruzione possa innalzarsi e competere a livelli europei. Questo ci si può aspettare da un Ministro dell'istruzione attento e responsabile; questo ci si può aspettare da un Governo credibile. Tutto questo purtroppo non è accaduto ed è sotto gli occhi di tutti, mentre è accaduto esattamente il contrario. questi insegnanti, che legittimamente speravano e continuavano ad avere diritto ad un posto di lavoro certo e stabile: per noi dell'Italia dei Valori costituiscono un grande patrimonio di cui il Paese non può fare a meno. Siamo in presenza del più grande licenziamento di massa dell'Italia repubblicana, che avrà conseguenze - anzi che sta avendo già conseguenze - dure e devastanti nelle Regioni del Meridione. Nessuno di noi, né il ministro Tremonti, ha il diritto di entrare così pesantemente nell'esistenza della gente, di condizionarla così tanto da azzerarne il futuro. Siamo fortemente convinti che bisogna investire nella scuola per dare al contrario agli studenti strumenti e preparazioni adeguate. Lo ha affermato magistralmente di recente anche il Capo dello Stato nel suo messaggio in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno scolastico. Riformare si può e si deve, ma con giudizio, signora Ministro. Siamo convinti che occorra anche elevare la qualità dell'insegnamento, motivando gli insegnanti, offrendo loro sempre più risorse; questa è la nostra convinzione. signora Ministro, è una precondizione essenziale e necessaria per lo sviluppo di un popolo. Se non si riconosce la priorità della ricerca e dell'istruzione, non si potrà mai assicurare al nostro Paese un adeguato sviluppo. Noi dell'Italia dei Valori restiamo fortemente e quotidianamente al fianco dei docenti, dei dirigenti scolastici (che malgrado tutto saranno chiamati a garantire ove possibile il massimo della qualità didattica), del personale ATA (che a causa dei tagli è costretto ad operare in condizioni ormai impossibili), dei precari della scuola (a cui non è stato rinnovato il contratto dopo tanti e tanti anni di serio lavoro), degli studenti e dei genitori tutti; restiamo al fianco dei tanti che non vogliono rassegnarsi e che vogliono piuttosto battersi contro provvedimenti gravi e inaccettabili come quelli in questione e che ogni giorno ci proponete; restiamo al fianco dei tanti che non vogliono rassegnarsi. Lo abbiamo fatto con grande determinazione nelle piazze, nelle sedi dei provveditorati, nelle sedi degli uffici scolastici regionali, incontrando giorno dopo giorno tutti gli operatori. Le assicuro, signora Ministro, è un coro unanime; io sono stato in Sicilia e ho girato tutte le Province, giorno dopo giorno, cercando di raccogliere le istanze di tutti quegli operatori per poi trasferirle opportunamente nelle sedi istituzionali. Lei ricorderà, signora Ministro, quante volte io stesso, nella qualità di componente della Commissione istruzione, ho esternato queste preoccupazioni e i tanti disagi. Ma quante volte le abbiamo invocato di fare insieme questa riforma? Lei lo ricorderà bene, ogni volta che è stata nella nostra Commissione glielo abbiamo chiesto con grande forza. Siamo convinti che oggi il tema vero è che la scuola è diventata precaria, questo è il significato delle nostre parole. Operare tagli indiscriminati nel campo dell'istruzione equivale a rendere precario il futuro di una collettività. In altre parole, signora Ministro, se la scuola è precaria, lo saremo anche noi, lo saranno anche i nostri figli. La verità vera è che voi, signora Ministro, considerate le politiche culturali, le politiche legate alla scuola, all'università e alla ricerca come marginali rispetto a quelle economiche e di bilancio. L'istruzione è un bene pubblico, è un bene che appartiene a tutti. Nessuno può e deve arrogarsi il diritto di distruggere tutto ciò. È per questo che non lasceremo solo chi ha il coraggio di far sentire la propria voce, dimostrando così amore per la nostra scuola e senso di responsabilità; quell'amore e quel senso di responsabilità che vediamo invece completamente assenti nell'azione di questo Governo. La scuola va salvata, signora Ministro, e per far ciò occorre prima di ogni cosa crederci e poi ancora l'impegno e la consapevolezza di tutti. Assumetevi la responsabilità di quello che state producendo nei confronti della scuola, nei confronti dei tanti professori, nei confronti del personale ATA, nei confronti degli alunni e dei genitori.

vi è sempre una notevole fatica a distinguere il suo pensiero e gli obiettivi tra quello che ascoltiamo e leggiamo nei dibattiti televisivi o sulla stampa e quanto poi nella nostra quotidiana attività parlamentare ritroviamo nei provvedimenti o nelle risorse destinate nei capitoli di bilancio di riferimento. Vorrei allora proporle alcune delle domande che le famiglie, i docenti, gli studenti le rivolgerebbero se lei avesse l'opportunità di entrare in una scuola normale domani mattina. Signora Ministro, non quale risposta normativa, ma rispetto alle bocciature che lei ha subìto da TAR e Consiglio di Stato, che cosa ha da dire a studenti e famiglie dal momento che nelle classi successive alla prima superiore negli istituti tecnici e professionali ha mantenuto i programmi e diminuito le ore di lezione? Quando pensa alla scelta politica della Germania del cancelliere Merkel di investire sul sapere 10 miliardi di euro, ritiene che quel Governo sprechi risorse, visto quello che dichiara sulla scuola italiana, o investa invece in speranza e futuro e dia possibilità ai suoi giovani di essere più competitivi nel mondo globale della conoscenza? Quella generazione di giovani capaci e meritevoli che lei di fatto esclude in questi cinque anni dalla carriera di insegnante. Si continua a sentire anche oggi l'ipocrisia della lezione sul merito, si continua a chiedere così tanto alla scuola, a volte troppo (l'insegnante che sostiene la famiglia, l'insegnante psicologo) e a chi insegna riconosciamo così poco, anche e soprattutto economicamente. Lei ci ha inondato di pagine, discorsi, norme sul merito con l'introduzione di meccanismi retributivi che dovrebbero prevedere insegnanti migliori, tranne poi cancellare nell'ultima manovra finanziaria il comma 9 dell'articolo 64 della legge n. 133 del 2008 fino alla fine del 2012. Abbiamo capito bene: fino alla fine del 2012! signora Ministro, penso che la maggior parte del mondo della scuola non voglia attendere né così a lungo, né questo Governo, né lei come Ministro. Si è mai chiesto, signora Ministro, perché, dopo l'approvazione in 7a Commissione del decreto-legge n. 112, con il taglio di 8 miliardi di euro nel luglio del 2008, non solo il Capogruppo del Partito Democratico, ma il capogruppo del PdL Asciutti e quello della Lega Pittoni chiesero l'audizione urgente del ministro Tremonti per i tagli eccessivi, come risulta agli atti? Secondo lei, signora Ministro, la chiesero per motivi ideologici, come ha detto pochi minuti fa, o perché volevano parlare col proprietario della borsa? Ministro, almeno con la legge Moratti-Bertagna si era di fronte a un progetto, discutibile ma che imponeva un confronto. Grazie a quel famoso articolo 64 della legge n. 133 del 2008 il riordino delle scuole superiori si è potuto ottenere solo con un parere in Commissione a mio parere, è una vergogna per il Parlamento), senza possibilità di emendamenti, di discussione in Aula, con i quadri orari che sono stati presentati senza i programmi che sarebbero arrivati quattro mesi dopo: l'importante è stato risparmiare sulla scuola pubblica. Tutte le ore disciplinari sono state ricondotte a frazioni di 18 per non avere nessuno «spreco», con ore a disposizione, conseguendo così, in taluni casi, l'assurdità della riduzione delle ore di inglese da quattro a tre perché 4 - lei ci insegna - non è sottomultiplo di 18. In questo lei ha veramente valorizzato l'inglese! Dalla sua relazione, signora Ministro, emerge un'unica certezza: abbiamo una scuola più povera e anche una scuola più parcellizzata e più divisa, non per quel federalismo proclamato ma mai attuato, ma una scuola dove i più problematici, i diseredati, i disabili da oggi sono anche un po' più soli. E dicendo grazie, nonostante tutto, alla professionalità e all'impegno di tanti insegnanti, questa sua scuola che esclude e abbandona non ci piace.

voglio ringraziare non tanto per quanto lei ha detto in quest'Aula ma soprattutto per quanto ha fatto. Le cose che ha detto noi della maggioranza le conoscevamo già; i colleghi dell'opposizione le conoscevano già, ma fanno finta di non conoscerle. Allora, perché la voglio ringraziare? Perché, a mio avviso, gli strali dell'opposizione si vanno sempre più rafforzando contro di lei. Perché lei, per quanto giovane, nel

e non si rendono neanche conto che, per la verità, più che non fare una riforma senza soldi, bisogna spendere meglio i soldi che si hanno.

e questo è un disagio che paga il Paese: bisognerà trovare una soluzione. Lei ha provato a indicarcela, peraltro parlando

nuove norme. L'avvio dell'anno scolastico è ritualmente un passaggio delicato, stante l'esigenza di trovare nuovi assetti nell'organizzazione scolastica e considerato che in essa è coinvolto tutto il Paese, tra studenti, famiglie, docenti, personale non insegnante. Quest'anno in particolare è stato un avvio denso di novità, tenuto conto dell'entrata in vigore delle nuove norme sul secondo ciclo esaminate a lungo dal Parlamento. Si tratta di una riforma perfettamente in linea con l'obiettivo del Governo di restituire serietà alla scuola, senza tuttavia gravare sugli studenti in termini di eccessivo numero di ore e di materie. Le polemiche che hanno investito l'inizio del nuovo anno risentono senza dubbio dell'impatto della riforma, che deve avere il tempo di essere monitorata a regime, una volta consolidata sull'intero quinquennio. Nessuno infatti certamente perfetta: la si potrà modificare una volta che l'avremo monitorata a regime e avremo verificato gli effetti che essa avrà prodotto. Peraltro, va sottolineato che le iscrizioni hanno premiato le novità e, per la prima volta, hanno valorizzato il settore tecnico-scientifico. Dai dati del Ministero emerge infatti che per il liceo scientifico, opzione scienze applicate (quella senza il latino), e per il riordino dei tecnici (in particolare nel settore tecnologico) l'aumento delle iscrizioni rispetto al precedente anno è dell'1,7 Inoltre, mi piace ricordare che, tra le principali innovazioni della riforma, hanno riscontrato il favore degli utenti il liceo linguistico (+1,3 per cento), il liceo delle scienze umane con opzione economica (+1,6 licei coreutici, le cui sezioni attivate sono al completo. Sempre nel merito del riordino del secondo ciclo, faccio notare che le recenti pronunce del giudice amministrativo - questo anche per rispondere prima che lo faccia lei - non hanno affatto inficiato il nuovo sistema imponendo una revisione di tutte le classi 2a, 3a e 4a degli istituti tecnici, come da taluni polemicamente sostenuto sull'avvio dell'anno scolastico: anzi, il Ministero ha chiarito che si tratta esclusivamente di tener conto del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella determinazione degli organici di riferimento della sentenza. Quanto alle presunte riduzioni di posti per il personale docente, occorre segnalare che il Governo era già intervenuto per ridurre l'impatto sui precari, introducendo ad esempio il meccanismo della precedenza nell'assegnazione delle supplenze temporanee, inizialmente previsto solo per l'anno 2009-2010 dal decreto-legge n. 134 del 2009. Rammento che in tale occasione, in qualità di relatore, avevo proposto che la misura fosse estesa anche al 2010-2011, proponendo un emendamento poi trasformato in ordine del giorno e recepito dal Governo. Adempiendo all'impegno assunto dinanzi al Parlamento, l'Esecutivo ha quindi provveduto a prorogare l'efficacia di quella disposizione attraverso il decreto-legge Si tratta evidentemente di un segnale di attenzione tanto della maggioranza, che ha sollecitato l'estensione delle norme al successivo anno scolastico, quanto dell'Esecutivo che si è fatto carico dell'attuazione concreta della disposizione al fine di garantire un margine a tali categorie di insegnanti. Per questi ultimi, peraltro, c'è comunque la possibilità di partecipare a progetti regionali, che offrono un altro sbocco lavorativo, seppure temporaneo. Quest'anno sono stati assunti 10.000 nuovi docenti e 6.500 nuove unità di personale va poi dimenticata l'approvazione definitiva del nuovo regolamento sulla formazione dei docenti, che è stato a lungo all'attenzione della Commissione per l'espressione del prescritto parere, mediante il quale si attiverà una nuova modalità di formazione parametrata alle reali necessità,

tanti edifici di civile abitazione, laddove usare il termine «civile» spesso è un eufemismo, vengono utilizzati per allocarvi le scuole, creando tra l'altro un meccanismo di spese eccessive ed anche inutili, anche questo uno spreco di risorse rispetto al quale dovremmo forse intervenire per tempo.

dovere. Lei ha dato una rappresentazione dell'avvio dell'anno scolastico che non corrisponde alla realtà. Nella realtà, nelle scuole, c'è una buona dose di caos, ma lei questo caos l'ha chiamato ordine, ed ha anche sostenuto che i tagli servono per una scuola migliore e per realizzare investimenti. Noi, sommessamente, vorremmo farle osservare che vediamo la realtà in modo diverso, e vogliamo dirlo alle famiglie italiane e agli studenti: vogliamo dire che il suo progetto di scuola e le misure che ha proposto sono parte consistente del fallimento politico e culturale del Governo di cui lei fa parte. Le chiedo che cosa vi sia di epocale - come lei le ha definite - in misure definite - in misure assunte esclusivamente per sostenere un taglio di 8 miliardi e mezzo di euro in tre anni. Ci spieghi in base a quale teoria pedagogica dovrebbe essere migliore e più meritocratica

di tantissime classi, decine e decine di migliaia di classi nel nostro Paese. Ci spieghi perché dovrebbe essere migliore una scuola dalla quale è destinato a scomparire uno dei tratti migliori della nostra tradizione, il tempo pieno, che non è il doposcuola, non è un tempo parcheggio per i bambini che non saprebbero altrimenti dove stare nel pomeriggio. Il tempo pieno è una modalità didattica più ricca, più coinvolgente, più produttiva di risultati: quello fatto di 40 ore con la compresenza degli insegnanti. Ecco perché le scuole che si sono attrezzate per questo e le famiglie che hanno potuto apprezzarne i vantaggi sono preoccupate dalla sua riduzione. Le cifre sul tempo pieno, quello vero, dicono che sono 70.000 gli alunni che ne sono rimasti esclusi, che sono 800 le classi in meno rispetto all'anno precedente e che se si fosse risposto positivamente alle nuove richieste, sarebbero state necessarie altre 2.000 nuove sezioni, naturalmente non concesse. Certo, dice il Governo, come si fa ad assicurare il tempo pieno se bisogna ridurre il numero degli insegnanti? Ma è questo il punto! Sembra incredibile, ma anche avere meno insegnanti di inglese, di informatica, oltre che di italiano, di storia, di musica, nella sua stravagante - me lo consenta teoria pedagogica, è considerato un fatto di qualità. Come lo è il dimezzamento dei laboratori, l'impossibilità di fatto di esercitare l'autonomia. È stato fatto un conto da una mamma: dalla scuola primaria alle superiori i nostri giovani studenti ed alunni È una scuola migliore quella che si svolge in edifici vecchi, malmessi, troppo spesso non sicuri, dove mancano le risorse anche per garantire l'igiene minima e la pulizia dei locali? Cento milioni sono una cifra davvero soltanto simbolica. Nella sua riforma "epocale" lei ha fortissimamente voluto il maestro unico, come ai tempi che furono. Ma lo sa, signora Ministro, che soltanto il 3 per cento delle famiglie lo ha scelto?

non si poteva e non si deve distruggere ciò che ha fatto diventare un segmento di eccellenza la nostra scuola primaria, frutto di anni di investimenti in risorse umane, in insegnanti di grande valore e competenza, in una didattica moderna che mette al centro la crescita dei bambini in una fase cruciale per la loro maturazione. Molti di quegli insegnanti, signora Ministro, oggi vogliono lasciare, abbandonare la scuola: vanno in prepensionamento. Si sentono demotivati, maltrattati anche, puniti dallo scarso riconoscimento del loro ruolo e della loro funzione formativa ed educativa. A lei sembra legittimo e normale che si licenzino decine di migliaia di insegnanti con anni e anni di servizio alle spalle, che hanno partecipato a corsi di formazione, di aggiornamento? Insegnanti espulsi nel nome di una migliore qualità della scuola! Lei ripete spesso - lo ha fatto anche oggi - che la scuola è stata considerata negli anni un ammortizzatore sociale. Ma lei, signora Ministro, confonde le cose: vi sono stati anni nei quali la scuola pubblica di qualità è stata la molla dell'emancipazione sociale, e per questa funzione - cioè la creazione di eguale cittadinanza - è stata al centro dell'attenzione della cultura, della ricerca pedagogica, delle istituzioni, della politica e quindi dei Governi. Ci ritroviamo a rimpiangere quegli anni fecondi alla luce della scarsa cura, perfino del disprezzo, che questo Governo manifesta verso la scuola pubblica. Purtroppo per il nostro Paese e per il futuro dei nostri giovani, tanto più rimpiangiamo quel tempo quanto più sarebbero necessari maggiore attenzione e maggiori investimenti per essere coerenti con la giusta strategia europea della costruzione della società e dell'economia della conoscenza. Con questo Governo siamo diventati il Paese che non dà il minimo contributo alla realizzazione di quella strategia. Ad esempio, avremo non meno, ma più dispersione scolastica. Inoltre quest'anno sono già alcune migliaia - lei non ne ha parlato, signora Ministro - i bambini in lista d'attesa per la scuola dell'infanzia: e sì che la nostra legge (ancora vigente) parla di generalizzazione della scuola dell'infanzia, il che significa che tutti i bambini ne hanno diritto. i bambini ne hanno diritto. E poi, non sappiamo ancora se per l'anno che è appena iniziato saranno attivate le sezioni primavera. L'Europa ci chiede di investire sull'educazione lungo tutto l'arco della vita, ma anche su questo si registrano disfunzioni e riduzioni di organico che portano ad avere nella scuola per adulti classi anche con sessanta studenti (sta succedendo a Firenze). E non ci dica, per favore, che occorre farsi carico tutti della crisi: nel luglio 2008, quando Tremonti e Berlusconi hanno deciso questi tagli, la crisi non si vedeva ancora all'orizzonte. E, comunque, ci spieghi perché altri Paesi, come la Germania o la Gran Bretagna, anche durante la crisi hanno consolidato ed accresciuto le risorse per l'istruzione e la formazione, mentre lei invece le ha drasticamente tagliate. Sappiamo tutti che nell'istruzione, nella formazione e nella ricerca sta la possibilità di sviluppo, di compatibilità e di dinamismo di una società. Altri Governi sono più conseguenti e più cooperativi rispetto all'obiettivo dell'Europa; noi no, ce ne allontaniamo. Come viene registrato dal rapporto OCSE, spendiamo per l'istruzione il 4,5 per cento del PIL. Siamo agli ultimi posti, insieme con la Slovacchia: la media europea è del 5,7 Quei tagli corrispondono ad una convinzione, signora Ministro, e ad un progetto: indebolire la scuola pubblica per realizzare risparmi e per dare più forza alle scuole private, quelle fatte per i ceti più abbienti e in grado di formare le classi dirigenti. Altro che scuola come ascensore sociale! Con le sue cosiddette riforme epocali, la mobilità sociale nel nostro Paese, già molto scarsa, si ridurrà ancora di più. Avete perfino ridotto l'obbligo scolastico, consentendo l'apprendistato a quindici anni. La verità è che la destra sta disegnando una scuola meno inclusiva e che dà meno opportunità ai giovani. rimproveriamo, signora Ministro, di non tutelare i settori sui quali il suo Dicastero ha la competenza, settori fondamentali per lo sviluppo sociale, civile ed economico del Paese. Le rimproveriamo di accettare senza condizioni di essere il braccio operativo del Ministro dell'economia. Oggi, purtroppo, ce lo ha confermato. signora Ministro, nel nostro programma elettorale noi abbiamo messo, come primo punto della riforma della scuola, la rivoluzione del merito. Io credo che la rivoluzione del merito sia la vera rivoluzione di cui abbia bisogno la scuola italiana. Sotto questo profilo e da questo punto di vista, io sono d'accordo con lei e sono d'accordo con l'operato svolto da lei e dal Ministro dell'economia, che la scuola italiana avesse bisogno di alcune razionalizzazioni. D'altro canto, non è lei il primo Ministro ad aver avviato queste razionalizzazioni; il ministro Moratti e poi, successivamente, anche il Governo di centrosinistra. Non dimentichiamo che i tagli agli organici vennero già attuati in misura significativa nella passata legislatura.

è la previsione che una parte dei risparmi derivanti dai tagli di organico sia destinata alla valorizzazione del merito. Ed è proprio su questo punto che io, signora Ministro, le chiedo di proseguire in quella logica meritocratica che è alla base del programma elettorale ed anche delle sue dichiarazioni programmatiche. Quel 30 doveva essere destinato a valorizzare la professionalità dei docenti, cioè a pagare di più gli insegnanti bravi. Lei aveva anche quantificato - se non ricordo male - una cifra importante, qualcosa come 2 miliardi e 400 milioni di euro o qualcosa di simile. quindi di una cifra significativa, che avrebbe potuto e potrebbe, se utilizzata correttamente, rappresentare finalmente una boccata d'aria fresca per la nostra scuola, che è sempre stata molto egualitaria e non ha mai valorizzato chi è bravo, chi si aggiorna, chi fa il proprio dovere fino in fondo e chi ottiene risultati di qualità. Affermo con

Noi abbiamo realizzato una rivoluzione autenticamente meritocratica: per la prima volta nella pubblica amministrazione, con riferimento ai docenti universitari, gli scatti non sono più automatici, ma sono legati ai risultati raggiunti.

di introdurre criteri meritocratici nella formazione e selezione degli insegnanti, ma non hanno - a mio avviso - raggiunto quei risultati che probabilmente una seria riforma, come quella in discussione alla Camera dei deputati, potrebbe assicurare alla scuola italiana.

iniziare a pensare quante risorse vogliamo mettere sul tavolo per poter risolvere questo grande problema sociale. Quando si parla, infatti, di centinaia di migliaia di persone è evidente che non possiamo scherzare. Non possiamo congedare gli

I calcoli che fece l'economia - mi permetto di dirlo - erano chiaramente sbagliati, tant'è vero che gli esperti del suo Ministero li avevano contestati e credo che da questo punto di vista il costo dell'operazione sarebbe di qualche decina di milioni di euro per il meccanismo delle compensazioni,

perché hanno un significato molto preciso nel linguaggio parlamentare. La condizione era che nella prossima finanziaria gli stanziamenti per l'offerta formativa tornassero a crescere tornassero a crescere di qualche decina di milioni di euro. Non si tratta di cifre enormi perché il capitolo di spesa è relativamente modesto, ma è importante per alcuni settori strategici. Penso, per esempio, alla riforma che lei ha fatto dell'insegnamento dell'inglese nelle scuole elementari. È chiaro che se continuiamo a tagliare i soldi per la formazione di questi insegnanti che non conoscono la lingua inglese, prendiamo in giro le famiglie perché queste si attendono che nelle scuole elementari il bambino impari l'inglese quando, invece, si trova magari davanti un persona che, a parte qualche verbo e qualche sostantivo, non riesce a parlare in inglese di fronte al bambino.

i soldi a disposizione delle scuole sono molto limitati e credo che la funzionalità delle scuole debba essere sempre e comunque garantita. Vi è, infine, il tema dell'edilizia scolastica. Quando ero assessore provinciale a Milano feci feci fare uno studio sulla scuola intelligente e risultò che alcuni accorgimenti rendono molto più efficace l'insegnamento e l'apprendimento dei bambini.

ci ha detto e nel ricordare alcune cose che andrebbero fatte. La Presidenza ci ha consentito una bella occasione: partecipare all'inaugurazione dell'anno scolastico parlandone in però voluto ascoltare quanti ragazzi e quanti bambini il 15 settembre sono entrati in classe, se sono aumentati o diminuiti, quanti sono gli stranieri, cosa accade per le persone disabili

E perché mai impariamo a vivere facendo roccia e tutte quelle attività che sembrano paramilitari quando, invece, abbiamo bisogno di palestre, di educazione civica, di educazione fisica: bisogna far crescere nella competizione, ma in quella sportiva, che insegna anche a rispettarsi.

investire in infrastrutture, perché non pensa a un piano pluriennale straordinario di edilizia scolastica? Avemmo un grande Ministro che pensò così e realizzò per la sanità un programma decennale in sede di finanziaria.

perché la meritocrazia senza la democrazia diventa selezione. Ma selezione di chi? Una scuola che compito ha se non quello di non perdere nessun talento del Paese? Abbiamo bisogno di portare avanti tutti, al massimo delle capacità di ciascuno. È un loro diritto, ma è un diritto del Paese avere talenti, altrimenti lo sviluppo di questo Paese chi lo garantisce? Tutti gli altri Governi che hanno

Il «manteneteli ignoranti e saranno ubbidienti» è la cosa più drammatica in un sistema democratico, perché non ci sarà capacità critica. Noi non vogliamo che la pensino tutti come noi, ma che siano liberi di pensare.

tramite lei, purtroppo non abbia ancora detto al Paese che la scuola è il vero tesoro da far fruttare. Questa è una scuola povera di contenuti, di insegnanti e di fondi; una scuola povera che renderà povero il Paese.

anch'io vorrei partire da alcuni dati, non solo perché sono ingegnere, ma anche perché credo che i numeri rappresentino la maniera migliore

Grazie

Abbiamo avuto anche una contrazione delle classi (da 1.363 a 1.332); solo nell'ultimo anno sono diminuite di 22.

Grazie

una tenuta, un'uguaglianza**,** forse una leggera contrazione degli istituti tecnici e una forte flessione degli istituti professionali. Anche questo è un dato da tenere in considerazione, perché sulla scuola professionale, invece, io ritengo che si debbano fare investimenti e incentivazioni.

Grazie

giusto utilizzo delle risorse economiche per quanto riguarda la scuola.

Innanzitutto, abbiamo visto, e possiamo affermarlo con assoluta tranquillità e serenità, che i tagli ai docenti non hanno avuto alcun effetto negativo nella scuola, per quella che è stata la nostra esperienza. A meno che non si voglia ricordare in maniera nostalgica l'organizzazione per moduli che, peraltro,

viene avvertita la mancanza di un sistema nazionale di valutazione che fissi i saperi irrinunciabili attraverso obiettivi minimi ed inderogabili per ciascuna classe e per ciascuna disciplina. Con riferimento invece alla gestione educativa degli alunni mediante l'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse, si riscontrano con alcune difficoltà, per gli ostacoli dovuti spesso a scarsa considerazione della scuola da parte delle famiglie, che faticano a riconoscersi nel patto di corresponsabilità da poco introdotto,

Signora Presidente, signora Ministro, l'anno scolastico che è da poco iniziato

fatta l'Italia, bisognava fare gli italiani, e il compito sostanziale di fare gli italiani fu affidato alla scuola pubblica, che fu inventata per questo, con l'obiettivo di educare alla cittadinanza, non nell'ora dell'educazione civica, ma attraverso tutte le materie, come si diceva una volta, attraverso tutte le discipline. In particolare, il cittadino italiano sarebbe stato costruito attraverso la competenza del sapere leggere, scrivere e fare di conto, proprio per evolvere la capacità di esercizio consapevole dei diritti-doveri della cittadinanza.

attraverso l'introduzione e la quasi piena realizzazione del principio universale del diritto allo studio, e la sua estensione a un'età dello sviluppo del bambino e dell'adolescente sempre più avanzata. viviamo tempi interessanti e lei, signora Ministro, si trova ad avere il privilegio e l'onere di fare il Ministro della scuola e dell'educazione in un'età molto interessante, perché è un'età di crisi ma, proprio per questo, è un'età che chiede alla politica

questo ministero è - glielo riconosco - assolvere al compito di elaborare un racconto dell'innovazione della scuola pubblica italiana, ma la forbice fra la realtà e questo racconto si è allargata sempre di più. Certo, è cominciato in salita. La realtà è è quella dei vincoli economici introdotti dal ministro Tremonti, che svolge in gran parte, lui stesso, il compito e il ruolo di Ministro dell'educazione, il suo tentativo di dare senso a questi tagli radicali è veramente impervio. È cominciato in salita - dicevo - nel primo decreto-legge di due anni e mezzo fa, allorché si tagliarono, tutti d'un colpo, 8 miliardi e mezzo di euro alla scuola. Il decreto, nel paragrafo fatidico che introduceva la figura del maestro unico, esordiva così: per le esigenze della razionalizzazione economica si introduce la figura del maestro unico. Non per esigenze pedagogiche. E il suo tentativo di dare senso a questa *gaffe* iniziale è un po' la cifra che ci porta ad oggi. Lei non ce la fa più, signora Ministro, a svolgere questo compito di dare senso ad una realtà che si sta sbriciolando. Non sto a ripetere la differenza fra il racconto e la realtà, che è stata ricordata dai miei colleghi,

non ci ha parlato della scuola, ci ha dato alcuni numeri. Lei stessa ci ha ricordato: "se guardiamo i numeri". No, proviamo a guardare le scuole, proviamo ad entrare davvero nelle classi scolastiche. Oggi le classi sono segnate da una grande sofferenza, da una grande difficoltà, ma soprattutto non sono accompagnate dalla domanda che noi, che abbiamo la responsabilità di riformare davvero la scuola, ci dobbiamo porre: che cos'è oggi la scuola? Quali sono i reali bisogni formativi dei bambini e degli adolescenti? Dobbiamo come chiave di lettura questa centralità della persona dello studente e non ricostruire il progetto della scuola a partire quasi esclusivamente da vincoli di sistema ed economici. Da che parte del mondo vuole stare l'Italia rispetto all'obiettivo non solo di Lisbona 2009, ma di Lisbona 2020? Oggi noi sappiamo che in tutti i Paesi del mondo conoscenza, democrazia, meritocrazia e sviluppo non possono che stare insieme. Il grande timore che in molti di noi, soprattutto nelle famiglie, soprattutto nella gente della scuola, ormai si sta affermando è che il futuro del nostro Paese non lo vedrà nel novero dei Paesi sviluppati, perché nella società della conoscenza non si tratta di produrre da parte di ciascun Paese

di un sostegno, perché tutti e ciascuno, i bambini e le bambine, possano immediatamente esprimere i loro meriti, le loro possibilità, le loro opportunità. mi lasci citare alcuni esempi paradigmatici delle difficoltà tecniche in cui ci troviamo. È stata fatta la riforma dell'ordinamento delle scuole superiori senza indicazioni:

di 12.000 posti per l'insegnamento dell'inglese nella scuola elementare contraddice la sua dichiarazione che la scuola che si apre quest'anno sia connotata da più inglese e da più scienza, da più matematica e da più tecnica. Ravvediamoci intanto che siamo in tempo, ma soprattutto costruiamo un progetto di scuola che sia davvero meritocratica. La scuola oggi è davvero in ginocchio. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore *(PdL)*. Signor Presidente, signora Ministro, senatrici, senatori, finalmente con il 1° settembre di quest'anno si è avviata l'attuazione della riforma del secondo ciclo di istruzione e formazione. Il complesso processo di riordino, a partire dalle prime classi, investe i percorsi della scuola secondaria superiore e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale. Il settore tecnico-scientifico è stato al centro delle principali innovazioni che, come dimostrano i dati sulle iscrizioni, hanno riscontrato il favore degli studenti e delle famiglie. L'aumento delle iscrizioni in tale settore è dell'1,7 per cento. Vengono incrementati gli orari della matematica, della fisica e delle scienze per irrobustire la componente scientifica nella preparazione degli studenti. È potenziato nel suo complesso lo studio delle lingue. La capacità di argomentare in forma scritta e orale e di saper leggere i testi complessi diventa un obiettivo comune a tutte le discipline. Nascono i nuovi istituti superiori post-secondari, cioè una nuova filiera non universitaria che dura due anni e che vede università, scuole e aziende protagoniste della formazione. È confermata con i fatti la linea del rigore: non si potranno superare i 50 giorni di assenza, pena la bocciatura. Aumentano le classi a tempo pieno, anche se qui qualche Cassandra preferirebbe il contrario, come è stato dispiace che non ci sia la collega Franco): quest'anno passeranno da 36.493 a 37.275. Mi dispiace per l'opposizione, ma aumentano. Sono stati assunto 10.000 docenti, come ricordava il Ministro, e 6.500 unità di personale ATA a tempo indeterminato. La legge finanziaria 2009-2011, tanto criticata dall'opposizione, comprende - è vero - tagli significativi e la riduzione del 10 per cento del personale insegnante su tre anni. Ebbene, è ora di ricordare che tale misura è coerente con gli impegni presi dagli ultimi due Governi per superare l'inefficienza della spesa pubblica. Come non ricordare il Quaderno bianco 2007 dei ministri Padoa-Schioppa e Fioroni che invito l'opposizione di oggi a rileggere perché ne ha bisogno, perché l'ha dimenticato. Grazie al ministro Gelmini andremo finalmente a riallinearci all'Europa sul numero di studenti per insegnante. Va ricordato che prima della riforma, ad esempio, il numero di insegnanti per 100 studenti nella scuola primaria era di 9,4 contro i 6,2 della media OCSE; nella secondaria di primo grado 9,7 contro 7,5; nella secondaria di secondo grado 9,1 contro 8. In tutti i tre livelli avevamo numeri superiori. Le ore di istruzione per la primaria 990 contro 796; per la secondaria di primo grado 1.089 contro 933; per la secondaria di secondo grado 1.089 contro 971.

L'elevato rapporto insegnanti-studenti è in gran parte basato su scelte politiche fatte in passato sul discutibile presupposto che un maggior numero di insegnamenti e di ore d'insegnamento insieme ad un minor numero di alunni per classe portassero a un miglior risultato. Le indagini internazionali stanno a dimostrare che tutto ciò è poco rilevante, se non del tutto irrilevante. Infatti, l'indagine PISA (*Programme for international fa riferimento, ha dimostrato che gli studenti quindicenni italiani hanno livelli di conoscenza, sia nelle materie letterarie che in quelle scientifiche, tra i più bassi dei Paesi dell'OCSE, e ciò malgrado la spesa per studente sia tra le più alte in Europa. È indubbio quindi che le tante risorse non sono ben investite. Del resto, è pur vero che gli insegnanti fanno tutti lo stesso mestiere, ma è anche vero che non tutti lo fanno con la stessa preparazione, impegno e determinazione Fino ad oggi, purtroppo, essi hanno lavorato senza nessuna valutazione, e quindi senza nessuna differenziazione, sia di qualifica che di remunerazione. La domanda che ci dobbiamo fare tutti è: perché nella pubblica amministrazione c'è un sistema di valutazione a tre livelli, mentre per la pubblica istruzione non

«Per decenni questa Nazione è rimasta intrappolata negli stessi stanchi dibattiti che hanno paralizzato il progresso e perpetuato il declino educativo. Troppi nel mio partito si sono opposti all'idea di compensare con incentivi economici l'eccellenza nell'insegnamento, anche se sappiamo bene che questi incentivi potrebbero produrre miglioramenti sostanziali.

e una accurata valutazione (...). Io sono assolutamente contrario a un sistema che premi l'insuccesso ed eviti che le persone siano responsabili delle loro azioni. La posta in gioco è troppo alta. Quando si tratta degli insegnanti dei nostri figli e della scuola in cui insegnano dobbiamo pretendere il meglio». Ebbene, valutare gli insegnanti e premiare i migliori: è la dichiarazione di un democratico, ma purtroppo non di un democratico italiano. Si tratta del presidente degli Stati Uniti d'America Del resto, signor Presidente, questa sinistra è rimasta ancorata alla protesta demagogica della scuola assistenzialista, della scuola di Stato a tutti i costi, alle rumorose e scomposte manifestazioni di oggi.

e purtroppo non riesce a districarsi da queste maglie. Proprio questa parte dell'opposizione è ancora convinta che la scuola sia un servizio utile per creare cattedre e posti di lavoro per docenti e personale, più che per istruire ed educare gli studenti. bisogna avere il coraggio di girare pagina. È ciò che ha fatto e sta facendo il ministro Gelmini, che personalmente ringrazio, e con lei il Governo e la maggioranza tutta, che dice no a una scuola intesa come una sorta di grande ammortizzatore sociale in cui immettere legioni di precari trasformati in maestri e professori, creando in questo modo costi insopportabili a scapito degli investimenti e della didattica. La scuola - di questo invece noi siamo convinti - deve essere un luogo dove si comunicano e si insegnano conoscenze e competenze, ma anche finalità e obiettivi; un luogo in cui il docente si riconosce nella sua missione di educatore, nella sua funzione di portatore di valori comuni e condivisi, oltre che di maestro istruttore o docente di contenuti didattici. La scuola, infine, come palestra di esperienza e di vita. È questa la sfida. È questa la prova, il salto che ci coinvolge tutti, genitori, insegnanti, istituzioni: offrire ai nostri ragazzi una scuola più qualificata ed efficiente, ma al tempo stesso più esigente. Restituire ai docenti, spesso demotivati e resi scettici da troppe frustrazioni, il prestigio e l'autorevolezza del loro ruolo. Dare certezze e serenità alle famiglie. È nel rapporto interattivo tra insegnanti, scuola e famiglia che lievita e matura la trasmissione di quei valori che corrispondono alla natura più profonda della persona. È vero, infatti, che i valori danno appartenenza, identità e passione, ma esigono anche rispetto. E il primo di tutti i valori è il rispetto di sé e degli altri. Il rispetto nasce dalla consapevolezza che esiste un valore intangibile che è la dignità di ciascuno come persona, e quindi la dignità di tutti, nessuno escluso. Tutto ciò, però, richiede alla scuola un *surplus*: quello di educare istruendo. Educare istruendo è un'aggiunta di responsabilità dell'adulto persona come docente, dell'adulto persona come genitore, dell'adulto persona come cittadino impegnato nella politica e nella società civile. io credo che si possa educare istruendo solo se come genitori, insegnanti e cittadini si danno esempi di vita e si è testimoni sui posti di lavoro, nelle istituzioni e anche nelle Aule parlamentari di ciò che si trasmette. Signora Ministro, vada avanti con le riforme necessarie: noi siamo con lei e stia sicura che anche l'intero Paese è con lei e con noi.

Ora, vorrei che lei non ci portasse solo dati e statistiche, anche se mi rendo conto che il suo ruolo oggettivamente deve poggiare su questo, così come le sue dichiarazioni. Allora, cominciando

del tutto impossibile provvedere alla sostituzione dei docenti assenti anche per un solo giorno. Questo è il quadro. Mi parlano di disparità tra classi dello stesso istituto.

Ogni volta che i bambini sono suddivisi tra le classi per la mancata sostituzione dell'insegnante assente si impedisce il regolare svolgimento della didattica sia nella classe scoperta, sia in quelle che accolgono i gruppi di bambini smistati. smistati. Sono problemi concreti, non legati ad una visione ideologica. Ed ancora, si rischia di riprendere la didattica trasmissiva, quella del dettato, del copiare, e di togliere ogni spazio alla creatività. Per non parlare della scuola media superiore, della scuola secondaria di secondo grado,

la dispersione scolastica. Attendiamo ancora i decreti relativi all'articolazione delle cattedre, ai criteri generali per l'insegnamento

un solo pensiero, una sola idea sui grandi obiettivi formativi per migliorare la nostra convivenza e su cui orientare i formatori. Niente sulla devianza minorile, dimenticando che la scuola non è fine a se stessa, ma strumento per trasformare in futuro reale le ansie e le speranze di una comunità nazionale. Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, ho chiesto al Gruppo PD della 7a Commissione di concedermi alcuni minuti per poter affrontare un segmento specifico del sistema scolastico pubblico italiano: le scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue nel Friuli-Venezia Giulia. Si tratta di scuole riconosciute, come d'altronde quelle italiane in Slovenia e Croazia, da accordi internazionali e regolate dalla normativa nazionale in materia di istruzione e da alcune leggi specifiche, ultima delle quali la legge n. («Norme a tutela della minoranza linguistica slovena»). Stiamo parlando di una realtà significativa, che rappresenta un valore aggiunto non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale. Alcuni dati per l'anno scolastico 2009-2010: 4.040 alunni, 480 docenti, 78 scuole tra scuole d'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. Si tratta, come potete vedere, di una realtà vivace e complessa che negli ultimi anni sta crescendo numericamente, anche grazie all'apporto di alunni provenienti da famiglie mistilingui o italiane che sono consapevoli dell'utilità di conoscere le due lingue del territorio. Anche queste scuole hanno iniziato il corrente anno scolastico con notevoli sofferenze: le difficoltà presenti nelle scuole italiane in seguito alle riforme approvate in questa legislatura e soprattutto ai tagli operati sono in qualche misura qui potenziate, visto che parliamo di un sistema con taluni aspetti specifici. Siamo pienamente convinti che la scuola italiana nel suo complesso abbia bisogno di cambiamento, di innovazione e di riforme; pensiamo però che esse non possano non tenere conto degli aspetti particolari delle scuole slovene nel Friuli-Venezia Giulia: il numero mediamente più basso di allievi, il maggior numero di ore di insegnamento, la necessaria dispersione di plessi scolastici localizzati nei diversi Comuni in cui vive tradizionalmente la minoranza slovena. È necessario perciò che le diverse riforme e gli interventi normativi e regolamentari non impoveriscano questo sistema e, soprattutto, non diminuiscano l'indispensabile offerta formativa; si tratta cioè di salvaguardare il diritto all'istruzione nella propria madrelingua, uno dei diritti fondamentali delle minoranze linguistiche, sancito anche da convenzioni internazionali. È per illustrarle tutto ciò che più volte ho fatto richiesta a lei, signora Ministro, di un incontro con i rappresentanti della comunità slovena. È da due anni che aspetto una sua risposta, salvo un cenno di promessa a fine luglio. Le si chiedono solamente la dovuta attenzione e la necessaria sensibilità verso questi temi. Per poter avere una visione più completa di tale problematica, sarebbe forse anche utile per lei visitare le scuole della minoranza italiana in Slovenia e Croazia.

su questo avvio dell'anno scolastico, in cui già si è avuta conferma, in alcuni casi anche in modo drammatico, di una istituzione scuola che fa fatica a stare al passo con i tempi e con l'Europa e, talvolta, fa fatica anche semplicemente a sopravvivere. Lei ci ha parlato con grande buona volontà, signora Ministro, della sua riforma, dell'istruzione secondaria, del riordino del sistema scolastico, dello sfoltimento degli indirizzi e dei risparmi di spesa. Ma per fare una riforma, signora Ministro, non basta solo tagliare le spese: occorre dare un'anima al rinnovamento legislativo, metterci dentro un'idea di sviluppo, di civiltà, di crescita formativa e di futuro. questa sembra una formula retorica, ma è la pura verità. Essa assume quindi un forte carattere sociale e culturale per il futuro del Paese. Se non si investe sui saperi, sulla ricerca e sull'università, non si investe sul futuro della nostra comunità nazionale. Centrare invece tutto sui risparmi, sulla lotta agli sprechi, sui tagli di personale (comprensibili) e sulle risorse rischia di compromettere seriamente i migliori propositi. Se, ad esempio, si accetta di tagliare in soli due anni più di 17.000 cattedre è chiaro che il futuro dei nostri giovani è solo quello di una riduzione delle ore settimanali di studio

si chiudono i laboratori, si sovraffollano le classi e si fa una politica di intervento solo ragionieristica? A distanza di due anni dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 112

87.000 cattedre e 44.000 posti di personale ATA), gli effetti sono sotto gli occhi dell'opinione pubblica perché gli esiti che si sono determinati sul nostro sistema di istruzione sono davvero pesanti. Si tratta di freddi dati numerici, ognuno dei quali però rappresenta una storia di vita vissuta da migliaia di cittadini e dalle loro famiglie. Non si può sfuggire poi alla drammatica cronaca quotidiana in cui si assiste all'elenco di un'infinità di disservizi, di problemi irrisolti, ma anche di casi umani di disperazione. È doveroso, ad esempio, ricordare in quest'Aula il tentativo di suicidio intentato solo ieri da un collaboratore scolastico precario di 51 anni a Palermo, il quale, dopo aver appreso che quest'anno non avrà alcun incarico perché il suo posto è stato tagliato, ha tentato

perché la prescrizione vincolante per legge imporrebbe di avere al massimo 25 alunni per classe per ragioni igienico-sanitarie, ma anche per ragioni di protezione civile.

Occorre, quindi, vedere con occhi diversi la quantità di risorse destinate alla formazione che solo così appariranno per quello che devono essere: vettori di qualità, di formazione dei cittadini da parte di istituzioni pubbliche che credono nel loro personale, che lo considerano una risorsa, un bene da valorizzare in vista del perseguimento di un bene pubblico essenziale come la scuola e la formazione, e non solo come una mera voce di spesa. Credo che in questo campo abbiamo subito troppo l'autorevolezza e la forza politica del Ministero dell'economia C'è bisogno di più scuola, di una scuola migliore. La riduzione del tempo scuola è sbagliata proprio perché va nella direzione opposta a quella in cui si muovono i Paesi europei più avanzati. Infatti, se è vero che diminuiscono i tempi della lezione frontale, è altrettanto vero che si allargano gli aspetti della nuova offerta formativa. anche dal senatore Valditara - che gli insegnanti italiani sono quelli meno pagati e i più anziani d'Europa, se poi si espellono migliaia di giovani docenti e si cancellano gli scatti stipendiali. Come si pensa di migliorare la scuola italiana? Si può governare la scuola contro il personale docente?

Occorre quindi reperire nuove risorse, magari aggredendo l'evasione fiscale. Se non si affronta il problema della scuola con questo respiro, si rischia solo di aggravare i problemi, deprimere le aspettative del personale docente, aumentare la dispersione scolastica, incrementare lo stesso divario fra Nord e Sud del Paese, con le energie migliori frustrate e costrette all'emigrazione intellettuale. Signora Ministro, nel campo della scuola si rappresenta in modo plastico, ulteriormente, il divario tra Nord e Sud del Paese, che è un tema che sta molto a cuore a noi del Movimento per le Autonomie. In questo quadro, infatti, il Mezzogiorno sicuramente, le isole e le zone montane subiranno i colpi più forti. Si accresce, anche per questa via, il divario già profondo tra le zone sviluppate e le zone svantaggiate del nostro La tendenza a privilegiare scelte di riforma nel campo scolastico in relazione al bilancio dello Stato, più che a fondarle su considerazioni esclusivamente di tipo pedagogico, approfondisce il solco determinato da scelte di politica scolastica che tendono a deprimere sempre più i territori più deboli in termini di strutture e servizi. Il tempo pieno è sufficientemente sviluppato al Centro-Nord, mentre al Sud rappresenta una rara eccezione. Da più parti le valutazioni concordano nello stimare che i tagli operati dal piano scuola sono concentrati per circa per circa il 50 per cento tra la Sicilia e la Campania. Il Movimento per le Autonomie si sente parte integrante di un profondo disagio del Sud del nostro Paese, posto di fronte agli esiti spesso catastrofici di provvedimenti che in astratto appaiono condivisibili, ma che calati nelle singole realtà appaiono, come sono, risposte uguali per situazioni profondamente diseguali. Cara signora Ministro, questo è un tema che allude a quello del federalismo: regole astratte e di principio che non tengono conto delle diverse realtà del Paese rischiano di determinare gravi ingiustizie. I meccanismi della perequazione devono essere valutati con estrema cautela e intelligenza politica dal Governo. La qualità dell'offerta della scuola pubblica nel Mezzogiorno rischia di essere seriamente compromessa dall'entità dei tagli del personale della scuola, sia docente che tecnico e di supporto. Gli insegnanti di sostegno, il cui numero viene costantemente diminuito al sopraggiungere di ogni finanziaria da diversi anni a questa parte, sembrano quasi scomparire in Sicilia, compromettendo seriamente il diritto allo studio per gli studenti disabili nella Regione. Nel Mezzogiorno il complesso della riforma viene percepito come un'ingiustizia. Non è quindi un caso che proprio nelle Regioni meridionali si sia creato un vasto e trasversale movimento di opposizione

Il tema della scuola è decisivo per garantire, pur in condizioni che si fanno via via più difficili sul piano economico e finanziario, un equilibrato progresso culturale, sociale e unitario dell'intero Paese. La scuola, l'università e la ricerca rappresentano l'unica garanzia di successo non solo per la vita di tanti giovani, ma anche dell'intero Paese. Non ci può essere sviluppo e crescita certa laddove permane e si approfondisce un squilibrio nello sviluppo anche e soprattutto nei territori meridionali. Per questi motivi vi è bisogno di un sistema scolastico che non penalizzi ma, al contrario, metta al centro le Regioni del Mezzogiorno, garantendo la lotta a ogni spreco ma, allo stesso tempo, il diritto allo studio e alla sua qualità. In conclusione, signora Ministro, è certamente necessario riformare la scuola, come per altro verso l'università, ma è importante che ciò avvenga appunto secondo un progetto, con un'idea di sviluppo solidale del Paese, che restituisca capacità di sviluppo ed efficacia al sistema scolastico e formativo nazionale senza il quale è in discussione il futuro stesso della nostra comunità nazionale. signora Ministro, non le porrò le tante domande che vorrebbero farle i genitori, gli studenti e gli insegnanti che così numerosi ho incontrato da quando lei è Ministro dell'istruzione. Il poco tempo a disposizione mi costringe a limitarmi ad un unico quesito. Le chiedo, signora Ministro: se il ministro Tremonti non avesse quantificato il contributo richiesto al suo Ministero nella prima manovra del Governo, prima che lei definisse le sue cosiddette riforme, avrebbe scelto le medesime misure e, soprattutto, gli stessi obiettivi? Io credo di no. Purtroppo, la sua informativa conferma ancora oggi la matrice tremontiana dell'operazione; mantiene un contenuto contabile fatto di numeri assoluti e relativi e conferma che il suo lavoro si esaurisce nel governare questi Ma dietro quei numeri ci sono bambini e bambine, ragazzi e ragazze cui devono essere garantiti i diritti; la sua rappresentazione tabellare senz'anima non tiene conto delle voci del Paese, che non è affatto tutto con lei come ha affermato il senatore Asciutti. Se sono solo lo 0,2 per cento le classi con 30 alunni, hanno scordato di raccontarle quali sono le percentuali di quelle che ne hanno 27-28 nella scuola primaria e nella scuola media. Signora Ministro, provi ad andare in una prima elementare fatta di 27-28 bambini, magari tre o quattro stranieri, senza intermediazione linguistica, oppure in presenza di un bambino con disabilità, senza copertura totale del sostegno. Provi, signora Ministro, a valutare quello che lei ha detto sugli insegnanti di sostegno: si è limitata ad affermare che sono aumentati di 2.500 unità. A mio avviso, un Ministro dell'istruzione si dovrebbe preoccupare di quanti sono gli alunni che, per poter vivere in modo proficuo il proprio percorso scolastico, hanno bisogno di un supporto. Ha proprio rovesciato il punto di vista. Vada a vedere, signora Ministro, come vengono non sostituiti gli insegnanti assenti: le classi vengono raccolte nelle palestre oppure sparpagliate in gruppi per l'istituto. Vada a vedere i laboratori di informatica, che non vengono aperti perché la mancanza delle compresenze impedisce di utilizzarli; vada a vedere i laboratori di musica dove le nomine nelle scuole medie non sono state attivate.

Avete azzerato i finanziamenti nell'edilizia scolastica e non avete neppure concesso una deroga al Patto di stabilità per poter intervenire in modo flessibile con questi interventi. Questi sono alcuni dei paradossi, signor Ministro, che vedrà, se vorrà fare un giro nelle scuole. E se lei ha dovuto sempre subire le decisioni del ministro Tremonti, cerchi di recuperare, perché non arriveremo sani al terzo anno di quella manovra. Faccia capire che è lei a capo del Dicastero più importante per le future generazioni e che non può chiudere gli occhi a fronte di tassi di disoccupazione giovanile ormai al 30 di un immobilismo sociale senza precedenti dal dopoguerra e di un aumento pericoloso degli abbandoni scolastici. Attiri l'attenzione del Governo dormiente verso il dramma sociale più evidente del nostro Paese: quello delle nuove generazioni. Credo, da quello che ha detto, che la risposta comunque alla mia domanda sia positiva, ossia insisterà in modo convinto nelle sue scelte, a prescindere dalle decisioni finanziarie. Non ci deve spiegare nulla. Non ci sono tabelle per capire ciò che, in fondo - lo dobbiamo ammettere - muove lei e la sua maggioranza: costruire un modello di scuola in cui chi è forte andrà avanti, chi è meno forte andrà avanti se potrà permettersi occasioni alternative nella scuola privata, e il resto si arrangi. Capiamo però anche perché le forze sociali ed economiche stanno predisponendo un nuovo patto sociale, alla stesura del quale il Governo non è stato invitato. Esse sono ben consapevoli di come scuola, università e ricerca siano strategici in un Paese che deve competere nell'era della conoscenza. Visto che poco avete ascoltato le minoranze e il Paese in piazza, speriamo che almeno loro abbiano la forza e gli strumenti per essere ascoltati.

L'altro giorno abbiamo saputo dal Presidente del Consiglio che la sua banalissima politica estera ha salvato il mondo. Da lei veniamo a sapere che sarà vinta la sfida dell'apertura dell'anno scolastico;

i temi del dissesto prodotto dalla legge finanziaria di Tremonti e dal suo procedere di conseguenza. Tagli, disoccupazione, precarietà; qualche collega ha parlato di licenziamenti di massa e, in effetti, in tre anni previsione è di 87.000 cattedre in meno e 44.000 soggetti in meno nel personale amministrativo. Si abbassa il numero delle ore settimanali, e questo è un artificio importante per dissimulare il calo dell'occupazione nella scuola. Le famose tre «i» (inglese, Internet ed impresa) rimangono ormai sospese: di inglese ce n'è meno di quello che doveva esserci; Internet, viene testimoniata da numerosi colleghi la riduzione degli insegnamenti di natura informatica e tecnologica; quanto all'impresa, sappiamo che in questo disgraziato Paese c'è solo un'impresa che riceve costantemente, anche negli ultimi mesi, aiuti diretti per il proprio sostentamento. Ogni tanto c'è qualche sprazzo di umorismo involontario: allènati o allenàti per la vita. Una cosa che soddisfa probabilmente la libido del ministro La Russa: avere a disposizione qualche ragazzotto per una specie di miniservizio militare di frodo. Ma forse la ragione dell'allenarsi per la vita dipende dal fatto che le statistiche dicono che ci sono 12.000 istituti a rischio dal punto di vista edilizio; probabilmente gli studenti devono essere allenati a fronteggiare

pieno. Gli studenti si alleneranno anche al fatto di avere meno insegnanti, meno insegnamento, meno formazione e meno cultura. Tutto ciò va di pari passo con una filosofia dichiarata apertamente da questo Governo: la svalutazione del valore dell'insegnamento. dell'insegnamento. Cari colleghi della maggioranza, voi dimenticate che gli insegnanti vanno pagati. Gli insegnanti italiani sono tra i meno pagati del mondo. C'è chi finisce l'insegnamento nella scuola media superiore non arrivando a 1.700 euro al mese. Poi ci tocca sentir parlare della dignità, della necessità di motivazione.

Come l'omino della favola veniva ricompensato dal suono della moneta, gli insegnanti precari, invece che da un giusto riconoscimento delle loro capacità professionali, vengono ricompensati dalla riconoscenza dei loro allievi, che sono grati loro perché si impegnano nell'insegnamento pur non pagati o scarsamente pagati.

che sono approvati dal vescovo, spesso bravissime e rispettabilissime persone, non attraversano un concorso pubblico e possono subentrare ai colleghi mancanti nei diversi insegnamenti. Immaginate il professore di religione, messo lì dal vescovo, che si ritrova a un certo punto ad insegnare Kant o l'illuminismo? In tale contesto, ogni tanto c'è qualche strappo di malagrazia. Se permette, signora Ministro, sono rimasto esterrefatto dal suo paragone espresso con la frase: tre mesi post-parto sono un privilegio; semplicemente perché lei, Ministra dell'istruzione, dotata di una provvigione significativa e di qualche agio materiale, si paragona al destino delle insegnanti che

soprattutto se uno sta nella dimensione scolastica di oggi, protestare è il minimo che si possa fare. Allora gli si dice: tu protesti, quindi fai politica; allora sei fuori dalla logica della scuola. Ho qui addirittura una inverosimile

prendendo sul serio il suo ruolo, io mi aspetterei seri provvedimenti nei confronti di una preside che può arrivare a delirare in questa maniera. Poi c'è la questione, la più importante di tutte, dei ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato che le hanno dato più volte torto. ricorsi - che non sto ad elencarle perché lei li conosce meglio di me - tutti relativi a irregolarità procedurali, all'ignoranza dei regolamenti e alla volontà di manifestare

la qualità degli insegnanti? Io vado per le vie brevi. Ho esperienza dell'argomento e so bene che è impossibile stabilire a priori un sistema per decidere se un professore sia bravo a insegnare Brunelleschi o l'entropia. La bravura e la qualità degli insegnanti saranno misurate (e di fatto lo sono già in parte) sulla base del criterio che viene premiato chi sta di più a scuola.

Si premia coloro che curano la biblioteca (che sono bravissime persone) e si premia chi porta in giro gli studenti alle mostre, ma il problema è misurare la qualità degli insegnanti. Questo è è un lavoro difficilissimo e presupporrebbe un'assoluta, condivisa buona fede nell'apprezzare i metodi della formazione e della trasmissione culturale, ma io non credo che da questa maggioranza, da questo Governo e da questo Ministero noi possiamo aspettare qualcosa su questo piano.

che cerca di fronteggiare il disinteresse della classe. Possono esservi classi interessate, per carità, ma possono esservi anche classi prive di interesse. Il vero maestro è quello che cerca di comunicare agli allievi il nucleo problematico della sua disciplina, che cerca di svegliare la curiosità, che cerca di seminare i dubbi nelle menti dei propri scolari cerca di dire ai propri scolari che lui non è la bocca della verità e che anche quello che lui dice può essere oggetto di dubbio e di critica. L'insegnamento di una disciplina è fondato soprattutto su questo esercizio sistematico dell'arte del dubbio. Lodoli spiega come si fa a gestire questo tipo di nucleo problematico di fronte a una classe che pensa al telefonino, oppure è semplicemente diseducata dalla società che gli sta intorno. Questo, infatti, è il nucleo, e vi sono classici che, recentemente, hanno parlato del fatto che

quale con questa riforma dell'istruzione voi passerete alla storia. Io ho il sospetto che voi passiate alla storia troppe volte: qualsiasi cosa facciate passate alla storia.

l'opposizione, in particolare il mio Gruppo dell'Italia dei Valori, di fronte a questa sorta di logica dell'annientamento, della rarefazione e dello svuotamento, si sente impegnata, più che mai, a sostenere le lotte che nel mondo della scuola i soggetti attivi, quelli che vogliono insegnare, che vogliono formare e che non vengono pagati abbastanza per farlo, si impegnano a fare. Il prossimo 8

qual è l'arte dell'insegnamento, che temo invece voi riduciate semplicemente ad un compito burocratico di conteggio contabile. Signor Presidente, signora Ministro, colleghi, si confrontano in Aula opinioni diverse, sembra che vediamo cose diverse, è come se parlassimo di un'Italia diversa. Dov'è la verità? In realtà abbiamo un'altra visione dei valori, degli obiettivi, degli strumenti: abbiamo un'altra visione politica. Lei, signora Ministro, ha parlato di inizio normale, regolare dell'anno scolastico. Se al posto mio oggi ci fosse però un insegnante, uno studente, un genitore, un dirigente scolastico della scuola italiana,

O non le parlerebbe piuttosto, come sta avvenendo in tutta Italia, delle migliaia di bambini esclusi dalla scuola dell'infanzia, che vuol dire un pezzo di vita in meno; del tempo pieno che non trovano più, delle pluriclassi aumentate sull'Appennino e sulle Alpi; della precarietà dell'insegnamento e dell'apprendimento; della qualità della scuola che viene inevitabilmente meno; del valore stesso della scuola pubblica, che è messo in discussione quando mancano le condizioni necessarie che fanno di una scuola una scuola, non un «taglia e cuci» di ore, un via vai di persone, una miseria di cui vergognarsi ogni giorno, senza progetto e senza sicurezza per il futuro? Non si fa una buona scuola se si vive nell'incertezza, nella sfiducia, nella preoccupazione. Una cosa così, come si fa a chiamarla riforma, e per di più organica? Signora Ministro, il senso della misura. Se fossero qui al posto mio, le racconterebbero dal vivo che cosa è diventata la scuola dopo i tagli della legge n. 133 del 2008, perché l'inizio è tutto lì; della sottrazione di risorse agli enti locali e alle Regioni. Di fronte a lei sta una scuola martoriata dai tagli, per usare le parole del segretario nazionale della CISL, Bonanni. In Turchia oggi - in questo grande Paese che vuole entrare in Europa - è in atto un piano nazionale denominato: «L'educazione toglie gli ostacoli». In Italia, invece, lei mette continuamente ostacoli all'educazione. Se fosse qui l'Italia che fa la scuola, che la ama e la vuole all'altezza del compito, oggi la inchioderebbe alle sue responsabilità politiche e con lei il Governo; e lo farebbe perfino con stupore e con sgomento - che sono anche i miei - perché nessuno nella scuola italiana avrebbe mai immaginato di poter essere considerato da voi un epigono, un residuo del '68, vista come un ammortizzatore sociale, com'è stato detto in quest'Aula la settimana scorsa dal Presidente del Consiglio, e come oggi anche lei ha ribadito. Ma non le viene il dubbio che il vostro approccio ideologico e miope stia determinando un danno mortale ad uno dei settori essenziali del Paese? Maneggiare con cura, signora Ministro, prendersi cura e, soprattutto, aggiornare la cultura politica, altrimenti rimaniamo inchiodati al passato. Ora sono qui io, con i colleghi parlamentari, a rappresentare il dolore, la rabbia, la passione di una scuola che non si arrende, che è determinata a non soccombere. Sono qui a rappresentare un Paese che ha bisogno di ben altra capacità di governo, che investa nell'istruzione (il primo obiettivo del sistema Paese), che preveda una programmazione seria dei pensionamenti e delle nuove assunzioni e una seria valorizzazione di chi è bravo, di chi lavora in zone difficili; interventi ben più seri sulla formazione dei docenti e sulla valutazione dei risultati (ci vuole ben altro che INVALSI e INDIRE) e un serio rapporto con le Regioni e con l'Europa. Sono qui a dirle che grande, signora Ministro, è la vostra responsabilità storica. Nel '62 il Governo di centrosinistra di allora aprì la scuola media a tutti; una rivoluzione culturale e sociale nel solco della Costituzione. Voi sarete ricordati per aver indebolito, negato il diritto fondamentale all'istruzione delle nuove generazioni, per avere sottratto loro opportunità anche nel confronto con i ragazzi del mondo. Ma lei pensa che i ragazzi italiani, con la sua scuola, saranno protagonisti attivi nel mondo di domani? La politica dell'istruzione, del resto, non è diversa da quella economica e sociale del Governo: la stessa inadeguatezza, la stessa assenza dell'idea di crescita. Signora Ministro, passerà il suo Governo; resterà una scuola italiana ferita e fiaccata, ma che non smetterà di credere nella sua missione, nonostante lei; resterà una scuola che crede nei resterà una scuola che crede nei ragazzi, in ogni area del Paese e di ogni condizione sociale, in quelli italiani e in quelli immigrati, rom compresi; che crede nella missione dell'insegnante e della sua professionalità, nel ruolo di dirigenti scolastici fedeli alla Repubblica, non al Ministro di turno e alla sua corte, fedeli al diritto. C'è un giudice a Berlino, signora Ministro: il Consiglio di Stato nei giorni scorsi ha registrato la vostra approssimazione, la vostra fretta, la vostra sciatteria. C'è una scuola che crede nei valori costituzionali, nella libertà, nella responsabilità, nella sua autonomia; una scuola che sa di essere fattore decisivo di uguaglianza, non di disuguaglianza, di coesione sociale e di convivenza civile, non di separazione dell'intero Paese dal Nord al Sud, senza le sceneggiate di Adro, della cui gravità lei all'inizio neppure si è resa conto. C'è una scuola che educa alla cittadinanza e alla democrazia, e per questo coltiverà sempre la speranza, nonostante questi giorni difficili e tristi. Signora Ministro, un *annus* *horribilis* è cominciato per la scuola italiana e il prossimo non sarà migliore, se continuerà così. Signor Presidente, signora Ministro, senatori e senatrici, desidero innanzitutto esprimere piena condivisione alla relazione del Ministro, che non è affatto generica come invece in qualche intervento da parte dell'opposizione - mi riferisco in particolare al senatore Zanda - si è sostenuto. Lei ha fatto chiarezza su molti importanti punti. La diminuzione del personale docente è stata quasi tutta assorbita dai pensionamenti, non ha dato grandi problemi. Non è vero che il numero degli insegnanti di sostegno sia diminuito: al contrario, è aumentato di 3.500 unità, e non sono poche. Non è vero che il numero degli alunni per classe sia così aumentato: lei ha citato un dato, ossia che le classi di 30 alunni sono lo 0,4 per cento del totale, che non è certamente un gran numero.

È stato varato il regolamento per la formazione iniziale degli insegnanti, che prevede tra l'altro accesso a numero chiuso e quindi la fine del fenomeno delle graduatorie e del precariato: si diventerà insegnanti dopo un percorso specifico di formazione ed un anno di tirocinio nelle classi. Si è dato un forte impulso alla informatizzazione della scuola e dei suoi insegnanti. Al riguardo mi permetto di ricordare quello che lei ha detto, signora Ministro. Alla fine di quest'anno scolastico saranno attive oltre 40.000 classi con la LIM, cioè la lavagna interattiva multimediale; un milione di studenti e 300.000 insegnanti saranno formati nell'utilizzo delle nuove tecnologie. La promozione della serietà degli studi si è manifestata in molti punti della sua azione legislativa in modo assolutamente meritorio. La linea di maggiore severità inaugurata col 5 in condotta con il rigore adottato nell'ammissione agli esami quest'anno registra anche una maggiore attenzione alle assenze: non si potrà superare il limite di 50 giorni di assenze se si vorrà essere promossi. Le prove di verifica alla fine della terza media introdotte dall'INVALSI saranno destinate ad ampliarsi alla scuola secondaria superiore e in prospettiva agli esami di maturità. Anche per gli insegnanti partiranno due importanti sperimentazioni per individuare criteri e metodologie per la valutazione degli insegnanti e delle scuole in vista dell'introduzione della carriera degli insegnanti. Sull'edilizia scolastica le segnalo, signora Ministro, una nostra inadempienza come Parlamento.

per ristrutturazioni in zone di particolare bisogno. Questo finanziamento era subordinato ad un parere delle Commissioni bilancio e cultura sia della Camera che del Senato; purtroppo, non si è ancora provveduto ad esprimere un parere al riguardo e credo che ci dobbiamo muovere con rapidità per sbloccare questo finanziamento.

primo luogo, l'apprezzamento per il pieno allineamento dell'azione del suo Ministero all'esigenza complessiva di austerità della spesa pubblica. Tale necessario ed indispensabile allineamento è ovviamente difficile, ma proprio perché difficile è meritorio e dimostra coraggio. Coraggio è la parola giusta. Il secondo ed ancora più importante apprezzamento è quello relativo alla profonda azione riformatrice posta in essere finora: riforma della scuola primaria, riforma della scuola secondaria, tra poco anche riforma dell'università; una rilevante azione riformatrice, in netta discontinuità con le dinamiche evolutive del passato. Lei fa onore con questa sua azione a quello che forse è l'impegno principale nei confronti dei cittadini del Governo Berlusconi: l'impegno del fare. L'adesione della sua azione al contesto generale della austerità ed alla finalità della diminuzione della spesa pubblica, i valori di meritocrazia e di serietà da lei vigorosamente promossi, il coraggio della sua azione riformatrice sono tutti contributi di grande importanza per la promozione della identità del centrodestra in questa legislatura. Vada davanti così, signora Ministro. Siamo al suo fianco per sostenerla nella sua azione!

Con lo stesso garbo cercherò di dire qualcosa che possa quanto più attaccarsi alla realtà, e quindi trascurerò alcune delle ... Stavo per Stavo per dire falsità, ma è troppo pesante: piuttosto qualcuna delle sue inesattezze, a cominciare dalla difesa del ministro Tremonti e dalla minimizzazione del tema delle risorse.

come diceva la collega Vittoria Franco, solo la Slovacchia ci batte. È poi vero che la spesa media annua per studente è di quasi 8.000 dollari, ma essa va principalmente a beneficio della scuola primaria e secondaria, a scapito dell'università: su questo fronte ci fermiamo a 8.600 dollari a studente, contro una media OCSE di quasi 13.000. Ho ascoltato con grande attenzione la sua relazione ne ho apprezzato alcuni passaggi e principi ispiratori; non posso tuttavia condividerla del tutto a causa della grave condizione in cui langue il sistema formativo italiano. tale condizione non è imputabile esclusivamente alle scelte del suo Dicastero, essendo frutto di errori e mancanze accumulate da molti differenti Governi; come negli anni precedenti, sarebbero stati necessari sforzi maggiori per iniziare a invertire questo *trend*. Mi chiedo come si possa non vedere che la scuola è ripartita qualche settimana fa esattamente come l'anno scorso, cioè tra caos e proteste. caos e proteste. La riduzione degli organici ha creato - bisogna ammetterlo - enormi difficoltà su larga scala, al Nord come al Sud. Ne sono conseguenza il sovraffollamento delle classi e il solito carosello di insegnanti. Nel sistema scolastico, prima che altrove, al tema dell'integrazione e al rispetto della disabilità occorre dedicare la massima attenzione; da qui bisogna partire per superare pregiudizi, disuguaglianze, ingiustizie: la scuola deve essere motore di eguaglianza e fattore di crescita. A ciò si aggiunga la mancanza di risorse per la didattica e l'amministrazione, nonché l'inadeguatezza di gran parte del nostro patrimonio edilizio scolastico, una vera e propria emergenza. Lei ha fatto

Urgenti appaiono dunque l'anagrafe scolastica e un serio piano d'investimenti. Vi è poi il dramma della riduzione del tempo-scuola, che comporta l'impoverimento l'impoverimento dell'offerta formativa e la contrazione dei posti di lavoro, aggravando la questione del precariato, che ha origini lontane e dimensioni oggi non più tollerabili. A questo proposito, con grande rispetto, vorrei richiamare l'attenzione del senatore Asciutti, che ha parlato di un'opposizione che ama la scuola ma che è impedita ad agire dai sindacati. Io non so se il senatore Asciutti sa

Per un momento, signora Ministro, lei mi ha deluso (per un momento solo) quando ha affrontato il tema del precariato parlando di ammortizzatori sociali nella scuola.

Sappiamo, come lei più volte ha ribadito, che gli stipendi per il personale rappresentano l'80 per cento di una spesa corrente in regolare aumento e conveniamo con lei che l'impiego delle risorse debba essere riequilibrato. Ciò tuttavia non giustifica il sacrificio di 140.000 precari, in strada da un giorno all'altro, equiparabile ad un licenziamento di massa. L'annuncio della possibilità di assorbimento entro sei o sette anni degli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ci appare di questo passo un traguardo eccessivamente ambizioso e comunque un tempo troppo lungo per le migliaia di precari. Quanto al reclutamento, esso va ancorato al merito, così come la stabilizzazione del personale va collegata alla formazione, e per elevare la qualità dell'insegnamento occorre motivare gli insegnanti. Io sono convinto che lei abbia il tatto per parlare con gli insegnanti, e non può non accorgersi dell'avvilimento che c'è. Non lo dico con spirito polemico, non è nel mio DNA, non può non rendersi conto dell'avvilimento che c'è nella maestra elementare che guadagna quattro soldi e non ha un minimo di rispetto. Non è questione di personalità o no, ma di essere messa ai margini dello Stato. Altra questione è la valorizzazione del personale: prendere atto del ruolo sociale vuol dire conferire dignità alla sua funzione, alla funzione dell'insegnante, perché no, un adeguato riconoscimento economico quantificabile attraverso il merito. Il Presidente della Repubblica, in un recente discorso, ha ricordato, accanto alle tante conquiste compiute dalla scuola in 150 anni, il grave ritardo da essa accumulato ed ha indicato, con chiarezza, le direttrici su cui orientare gli interventi: più qualità; un rapporto più stretto tra istruzione e mondo del lavoro; maggiore spazio alle competenze richieste nelle società contemporanee. Vogliamo quindi unirci all'appello del Capo dello Stato ed essere cassa di risonanza delle sue parole. Sebbene la crisi attuale e l'urgenza di ridurre il debito pubblico impongano sacrifici e rinunce, nella ripartizione delle risorse disponibili è doveroso riconoscere la priorità della ricerca e dell'istruzione. Apprezziamo il suo impegno in tal senso nel confronto con il ministro Tremonti e la invitiamo a continuare su questa strada. Siamo convinti che preparazione e formazione adeguate rappresentino la leva per uscire dalla crisi. Al contrario, questo Governo, con la sua politica di tagli - e qui la escludo, veramente senza riserve mentali - ha trasformato istruzione e ricerca nella cenerentola del Paese. E veniamo al tema dell'università. Il provvedimento attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento è sicuramente di grande importanza, in quanto tenta di realizzare una riforma da tempo e da più parti invocata. Sino ad oggi scelte discutibili ed onerose hanno prodotto effetti negativi, quali la proliferazione incontrollata di sedi e corsi, il disordine, l'inefficienza nella *governance* del sistema universitario e un generale abbassamento del livello qualitativo. Diversi sono i punti della riforma che condividiamo, signora Ministro: una *governance* caratterizzata da autonomia e responsabilità, criteri di reclutamento improntati alla meritocrazia, il tentativo di legare la carriera e la retribuzione dei docenti non ad automatismi, ma a produttività e qualità del lavoro. Ci chiediamo però come sia possibile fare tutto ciò senza risorse; una riforma così impegnativa richiede investimenti sostanziosi. Il Governo, al contrario, ha proceduto esclusivamente a tagli paralizzanti. Come di recente ha osservato anche il centro studi della Confindustria, il tasso di laureati tra i 25 e i 34 anni è troppo basso in Italia rispetto alla media europea,

Ciò finisce per incidere fortemente sulla competitività del sistema socio-economico, in quanto più bassi sono i numeri meno ricerca si produce divenendo inevitabilmente meno incisivi sul mercato globale. La scuola che lei sta disegnando, signora Ministro, non è ancora la scuola della valorizzazione dei talenti, non è motore di eguaglianza e fattore di crescita economico-sociale indispensabile allo sviluppo di un Paese come il nostro. Infine, non possiamo rassegnarci al fatto che un luogo - al riguardo vorrei che lei esprimesse condivisione, signora Ministro - deputato a coltivare e incoraggiare lo spirito civico e i sentimenti di solidarietà nazionale, particolarmente avvertiti nella ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, venga ricoperto di simboli che violano l'autonomia scolastica in spregio della Costituzione: simboli che rappresentano la volontà di frammentare il Paese e la sua identità. Non si può speculare sui bambini, sui ragazzi, sui giovani. *(Applausi dei non si ha senso della cultura, ovvero si ha solo il senso della cultura del voto*.* Da prefetto di Palermo spesso mi capitava di visitare le scuole del voto*.* Da prefetto di Palermo spesso mi capitava di visitare le scuole delle zone più sofferenti della Regione, zone in cui la diserzione scolastica raggiungeva tassi del 50 per cento, superiori anche ai tassi di disoccupazione. Lei non mi crede? La invito a fare un giro insieme verso Corleone e San Giuseppe Jato, se non mi crede. Come dicevo, spesso mi capitava di visitarle quelle scuole e là, signora Ministro, con grande sorpresa, ho trovato terreno fertile a tutti gli appelli alla legalità e alla speranza in un futuro migliore che rivolgevo alle nuove generazioni in veste di rappresentante del Governo. Quei giovani hanno fame di cambiamento, e il vero cambiamento passa proprio attraverso la scuola. Nella lotta contro le mafie non bastano le vittorie quotidiane che le forze dell'ordine mettono a segno contro latitanti e criminali: per ogni *boss* catturato, purtroppo, si contano decine di matricole pronte a prenderne il posto. La guerra contro le mafie, signora Ministro, si vince portando al Sud lavoro ed istruzione, ossia reali possibilità di riscatto personale, risposte concrete alla fame ed alla disperazione. Se lei vorrà perseguire questa missione e raggiungere un obiettivo si troverà davanti tantissime difficoltà, soprattutto da parte dei suoi alleati, signora Ministro, ma un'istruzione degna di tale nome è nelle sue mani, e noi confidiamo che lei potrà essere all'altezza. Signor Presidente, signora Ministro, colleghi senatori, l'ultimo rapporto OCSE sulla scuola evidenzia le clamorose anomalie del nostro Paese, ma commentatori interessati continuano a distorcere la realtà. Il tempo scuola dei nostri studenti è di gran lunga il più alto, con un valore nella scuola di base di circa 1.000 ore annue contro le 850 della media OCSE. Eppure, per qualcuno queste ore sono insufficienti. La disinformazione opera anche sulle risorse. Si fa notare l'incidenza della percentuale di spesa per la scuola sul prodotto interno lordo, ma è un confronto improponibile, avendo a che fare con troppe variabili. L'indicatore, invece chiarissimo, del costo per alunno viene trascurato. Per la cronaca, da noi è di 101.000 dollari, dalla prima elementare al diploma, contro una media OCSE di 94.500 dollari. Spendiamo quindi di più, anche se spesso male. In attesa, delle leggi attuative del federalismo fiscale (che riporteranno un po' di ordine anche nell'istruzione mettendo sotto controllo i conti), nell'immediato una partita possono giocarla le Regioni. Sulla base delle nuove norme fissate dallo Stato, i governi locali possono infatti legiferare non solo per l'organizzazione del servizio scolastico, vale a dire la dislocazione delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ma anche per la sua gestione, ovvero l'assegnazione del personale alle singole scuole (sulla base della dotazione organica assegnata dallo Stato) e la ripartizione alle scuole del territorio delle risorse finanziarie statali. Oggi, in assenza di leggi regionali per l'assegnazione del personale e dei fondi, lo Stato accredita direttamente alle scuole le risorse, sia di personale che finanziarie, necessarie per la gestione del servizio scolastico, con tutte le difficoltà aggiuntive che conosciamo. Ma c'è un'altra partita che possiamo - e dobbiamo - giocare. Provate a pensare se un domani, cercando un posto di lavoro pubblico, vi fosse la possibilità di essere valutati a parità di condizioni con chi proviene da altre Regioni. La domanda, per chi non conosce la realtà italica, apparirà strana. Ma il problema esiste. Di quest'estate l'ennesima conferma, con gli ultimi dati sulla maturità, che vedono le Regioni del Nord agli ultimi posti per percentuale di diplomati con il 100 e lode, mentre svettano per numero di eccellenti i licei di Reggio Calabria, Catania, Crotone, Cosenza. Conta poco se, al contrario, i test internazionali mettono ai primi posti gli studenti di altre realtà, non solo in Italia, ma addirittura a livello continentale. È a tutti evidente che, trattandosi di un problema di disomogeneità culturale tra le diverse aree del Paese, soluzioni facili non esistono. E, pur apprezzando i periodici tentativi ministeriali di varare piani per la qualità e il merito, crediamo sia arrivato il momento della concretezza. Il Sud non è tutto uguale. Piero Cipollone, presidente dell'INVALSI (Istituto che, pur con tutti i limiti dei *test*, ha il compito di individuare i punti deboli del nostro sistema formativo), segnala che l'Abruzzo ha valutazioni positive a livello della Valle d'Aosta e che Sardegna e Basilicata sono nella media nazionale. Il tutto per sostenere che «le Regioni indietro possono essere trainate da quelle vicine e riuscire a migliorarsi». Possiamo partire da qui. Nel progetto che abbiamo elaborato degli albi regionali per il reclutamento degli insegnanti, per assegnare il punteggio di base ai candidati alla docenza non si fa più riferimento (se non in misura ridotta, in una specie di «marcia di avvicinamento» all'auspicata abolizione del valore legale del titolo di studio) alla valutazione acquisita sul proprio territorio. Si dovrà scegliere una e una sola Regione nella quale eleggere il proprio domicilio professionale e sottoporsi a quello che abbiamo chiamato «test di preparazione», con cui si verificherà l'attitudine all'insegnamento e l'effettivo livello di preparazione dei candidati nelle singole materie. Il tutto - questo è il punto fondamentale - nella Regione di arrivo, a parità di condizioni con i candidati del posto. Il nuovo sistema da una parte eviterà che candidati valutati con «manica larga» in altre realtà possano scavalcare chi effettivamente merita; dall'altra metterà in "competizione" gli aspiranti all'insegnamento spingendoli a migliorarsi. Un candidato bravo, ma iscritto in una Regione dove i bravi sono tanti, sarà infatti spinto a iscriversi nella Regione vicina, che magari ha meno bravi e offre più opportunità di lavoro. A quel punto, però, gli iscritti in quella Regione avranno tutto l'interesse a darsi da fare per crescere professionalmente e non farsi sfuggire l'opportunità di conquistare la cattedra. Si attiverà cioè un percorso virtuoso, che può mettere fuori gioco il *business* dei titoli (brutta realtà in alcune Regioni) e la pantomima delle supervalutazioni, che per decenni ha relegato in fondo alle graduatorie diplomati e laureati delle Regioni padane, e non solo, bravi ma con valutazioni meno benevole rispetto ad altri territori. Il tutto nonostante la Costituzione, all'articolo 9, affermi che «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura» e tagliare il legame tra insegnanti e territorio significa uccidere la cultura. I disastri degli ultimi decenni al riguardo sono sotto gli occhi di tutti. La nostra non è una chiusura, ma il tentativo di ridare spazio a ciò che il territorio sa esprimere, che poi è la vera immensa ricchezza del nostro Paese. Un insegnante non trasmette solo con quello che dice, ma anche - e soprattutto - con la sua persona, per come è stata plasmata dal territorio. Oggi che crescere figli è diventato un lusso (per arrivare alla fine del mese spesso devono lavorare ambedue i genitori), le responsabilità della scuola nella trasmissione di cultura e valori locali sono cresciute in maniera esponenziale. E attenzione che la nostra proposta non contempla privilegi per gli insegnanti padani: non ne hanno bisogno. Gli albi regionali sono anche garanzia di continuità didattica, perché è vero che la maggior parte delle decine di migliaia di spostamenti di insegnanti che il sistema è costretto a subire ogni anno avviene a livello regionale, ma il problema è sempre lo stesso: docenti in buona misura originari delle Regioni meridionali, non avendo legami con il territorio e non potendo ottenere subito l'avvicinamento alla loro terra (laggiù le scuole sono perennemente ingolfate di personale), si spostano in zone meno disagiate. E la prima conseguenza è un *turnover* quasi del 100 per cento in montagna. Gli albi regionali favoriranno la presenza di insegnanti che, provenendo da quelle stesse zone, non hanno alcun motivo di scappare. È così che si garantisce la continuità didattica, non puntando la pistola alla tempia di chi non vede l'ora di andarsene, con provvedimenti coercitivi da sempre puntualmente aggirati. *(Applausi

parlamentare, un'occasione vera di confronto sulla scuola e non di ripetizione di *spot* già più volte presentati sulla stampa. Lei, invece, ci ha riproposto omissioni, silenzi, genericità che solo perché tante volte ripetute si può pensare che diventino credibili. I colleghi del Gruppo del PD hanno già parlato delle «voci della scuola» e hanno riportato qui quello che io non ho sentito nelle sue parole, cioè la scuola vera, quella che lei avrebbe potuto citare anche con grande orgoglio oltre che con problematicità, ad esempio citando le bellissime sperimentazioni di inserimento dei bambini stranieri nella nostra scuola, completamente ignorate, ovvero le esperienze positive di innovazione didattica che i nostri docenti stanno realizzando. Avrei voluto sentire nelle sue parole le voci dei dirigenti scolastici che affrontano reggenze molto pesanti, che dal Ministero devono ricevere mediamente 180.000 euro e non hanno più i soldi per fare nulla;

sono stati tagliati 132.000 posti di lavoro: si tratta di tagli e non di una razionalizzazione; è uno scardinamento di pezzi essenziali della qualità della scuola pubblica. È vero che lei parla dei pensionamenti; ma se però la FIAT avesse annunciato, ad esempio, di tagliare 132.000 posti di lavoro in tre anni, tutti avrebbero capito che quelli sono posti persi e che quei lavoratori non ci saranno più. Eppure lei lo nega. il tema del precariato non nasce da questo Governo, ma dobbiamo ricordare che negli ultimi dieci anni otto sono stati gli anni del Governo Berlusconi, e quindi qualche responsabilità su questo problema ci sarà pure! Inoltre, quando si è Ministri della Repubblica, non si risponde soltanto delle cose che sono state fatte, ma si affrontano i problemi esistenti; lei, invece, sta facendo di tutto per non affrontare questo problema, a cominciare dallo smantellamento del piano previsto dalla legge finanziaria del 2007 per assumere 150.000 persone in tre anni, cosa che avrebbe finalmente dato una sistemazione a quei precari che da anni si trovano in una condizione

destinate molte volte. Allora io le chiedo: ci può dire a che cosa sono destinate? Sono destinate - come io auspico - a recuperare il blocco degli scatti di anzianità? Ma per quanto durerà? Un anno, due anni, tre anni? E le ricadute, dato che il blocco è permanente per la scuola,

Innanzitutto, non è uno scandalo spendere per il personale, quando abbiamo una comunità educante: e gli educatori e gli insegnanti sono l'elemento fondamentale per un processo educativo.

in anno il suo peso all'interno della spesa pubblica (quest'anno, ricordiamocelo, il *deficit* pubblico è aumentato del 5,7 per cento). Ci vergogniamo, e riteniamo, però, di doverle chiedere una cosa. È vero che Tremonti sulla scuola ha voluto fare cassa

gli strumenti reali attraverso cui il Governo e anche lei state realizzando un disegno politico che, attraverso l'impoverimento e la dequalificazione della scuola pubblica, vuole spingere progressivamente

partitizzazione della scuola pubblica attraverso (la vicenda di Adro è gravissima) la marchiatura con segni di un partito politico; e io ritengo che lei abbia mostrato troppa tolleranza rispetto a questa vicenda, minimizzazione e reticenza, fino al silenzio assoluto nella sua relazione di oggi.

all'indomani della riforma della scuola superiore appena entrata in vigore. Questo primo bilancio dimostra che si sta andando nella giusta direzione: verso una profonda e radicale innovazione dell'intero sistema.

di una comunità sociale, una costante attenzione e preoccupazione da parte della politica e delle istituzioni. Ben vengano, dunque, informative come questa che si fondano su una conoscenza diretta della medesima realtà sulla quale le norme vanno ad incidere. In secondo luogo, la situazione in cui versa la scuola italiana è una situazione critica che affonda le sue origini nei decenni precedenti e che è attraversata da una serie di problematiche difficili da scardinare. Non è possibile, colleghi dell'opposizione, riferirsi a un periodo di dieci anni per poter dimostrare che c'è stata una prevalenza al Governo di una parte rispetto all'altra, invece la situazione fa riferimento a un contesto temporale ben più ampio che copre tutto l'arco della storia repubblicana. Il lavoro che si intende fare perciò è duro e complesso, ma ha un'ambizione grande: mettere fine, una volta per tutte, a questo stato di crisi; compiere una svolta che consenta un cambiamento radicale. Per rimettersi in carreggiata - questo è un fatto e non un'opinione - la scuola ha bisogno innanzitutto di razionalizzazione, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista strutturale. Specialmente nelle fasce più alte dell'istruzione: quelle più vicine alla realtà lavorativa e, quindi, determinanti nel rilancio dell'offerta formativa. In tal senso, il quadro tracciato oggi e determinato dall'introduzione della riforma mostra i primi segni soddisfacenti, in linea con i presupposti e gli obiettivi alla base del provvedimento, orientato verso una profonda innovazione che permette al nostro sistema di diventare più moderno e più competitivo. Due sono in particolare gli aspetti su cui, signora Ministro, vorrei soffermarmi, perché mi sembrano meritevoli di attenzione. Il primo riguarda uno dei mali che ha afflitto per decenni il sistema italiano e al quale, con questa riforma, si cerca finalmente di porre rimedio. Si tratta dell'incapacità da parte dell'universo scolastico di interpretare le richieste provenienti dal mondo del lavoro. In tal senso, la revisione degli ordinamenti avvicina la scuola italiana alle esigenze del mercato, alla crescente internazionalizzazione e alla richiesta di specifiche figure professionali. Il nuovo impianto ordinamentale degli istituti tecnici e professionali, dotato del grado di autonomia necessario per adattarsi a singoli contesti territoriali, rivaluta fortemente un settore in cui l'Italia è stata purtroppo carente negli ultimi decenni, e crea un'occasione di orientamento autentico nei confronti di quegli studenti che in questi anni hanno fatto fatica a canalizzare il loro talento. Signora Ministro, leggendo questa parte mi è venuto in mente come spesso la modernità coincida con la classicità, perché lei ha ripreso considerazioni e proposte presenti in una ipotesi di riforma che porta la firma di un grande pedagogista e di un grande storico, Galletti e Salvemini, e che formava

c'è un altro dato fondamentale da sottolineare, che non riguarda tanto gli aspetti tecnici del cambiamento in corso, quanto la portata e il valore politico di questo cambiamento. Per anni la scuola italiana è stata utilizzata come una sorta di ammortizzatore sociale: una riserva indefinita di posti di lavoro, moltiplicati all'occorrenza per stimolare il consenso elettorale. Anche questa, signora Ministro, è una pagina della nostra storia repubblicana con la quale dobbiamo fare i conti tutti con coraggio perché è la nostra storia, senza ritagliarci delle periodizzazioni di comodo. Seguendo questa logica irresponsabile sono stati assunti 200.000 precari e non è stato fatto nessun controllo sulla qualità degli insegnanti, affossando in questo modo il merito e mortificando gli eccellenti professori presenti nella scuola italiana stanchi di non veder riconosciuto e premiato il loro valore. È una storia che quelli della mia generazione conoscono perché l'hanno vissuta sulla loro pelle: sanno quale era la considerazione sociale dei professori dei loro licei, e sanno qual è la considerazione sociale dei professori dei loro figli. E' una situazione drammatica alla quale è necessario porre rimedio, e senza incidere su questo circolo vizioso porvi rimedio non è possibile. È inaccettabile - concordo pienamente con lei, signora Ministro che oggi l'unico meccanismo di progressione dello stipendio per gli insegnanti sia quello degli scatti di anzianità. logica, che offende il merito e premia l'egualitarismo, era possibile nel momento nel quale il riconoscimento sociale era selettivo. Non è accettabile nel momento nel quale quel riconoscimento è stato massacrato, perché oggi non si hanno né i soldi né la

È vero - come è stato detto, e ci tengo a ribadirlo - che sapere non significa necessariamente saper insegnare. Ma, a sua volta, saper insegnare non significa, colleghi della sinistra, cedere alle sirene del panpedagogismo degradando le singole discipline e i loro contenuti a meri accessori. È vero esattamente il contrario. Bisogna risollevare dunque il nostro sistema scolastico dallo stato di crisi nel quale lo hanno portato l'irresponsabile vendita di illusioni perpetrata fin troppo a lungo, e l'egualitarismo di matrice sessantottina secondo il quale tutti, i bravi, i meno bravi e coloro i quali bravi non sono, dovrebbero essere messi sempre sullo stesso piano. Signor Presidente, colleghi senatori, l'inversione di rotta era necessaria. Del resto, le grandi riforme si fanno proprio sfruttando le crisi, come accaduto anche altre volte nella storia d'Italia e per le migliori riforme che hanno riguardato la scuola. Andiamo a leggere a tal proposito gli atti sulla riforma Gentile. Al ministro Gelmini va dato atto di avere coraggiosamente intrapreso una strada difficile e piena di ostacoli, ma che va nella direzione giusta. Ciò è stato fatto *in primis* attraverso un'oculata razionalizzazione dei costi, grazie alla quale è stato possibile, tra l'altro, assumere quest'anno - riprendo dati riferiti dal Ministro - 10.000 nuovi docenti, 6.500 unità di personale e 170 dirigenti scolastici. Mettere ordine nelle voci di bilancio, nei capitoli di spesa e porre fine alle abitudini distorte del passato consente di fare di necessità virtù, a fronte di una congiuntura economica ed internazionale - un problema di cui tutti dovremmo farci carico - le cui ricadute non hanno risparmiato nessun settore, nemmeno quello dell'istruzione. Prendere a pretesto la dura responsabilità di far quadrare i conti per inscenare polemiche strumentali non fa onore a questa opposizione e a quella responsabilità che uno schieramento politico dovrebbe invece dimostrare, se vuole aspirare a governare il Paese. Il vero fulcro della riforma in atto è stato il taglio, quello sì, degli enormi sprechi accumulati nel tempo in direzione di una più razionale amministrazione delle risorse e dell'organizzazione del sistema scolastico; una razionalizzazione dettata dalla necessità di interrompere la crisi della scuola italiana, ma portata avanti tenendo conto che il sistema scolastico è fatto di persone in carne ed ossa, che vanno sempre tutelate e sostenute. Mi riferisco in particolare all'esercito dei precari, illusi da chi li ha assunti senza accertarsi prima dell'effettiva necessità e della sostenibilità economica di quelle assunzioni. Non riconoscere il nostro impegno in tal senso non soltanto non corrisponde alla realtà dei fatti, ma dimostra l'imbarazzo di chi ha contribuito ad affossare la scuola italiana e adesso non vuole dare a chi sta cercando di risollevarla il merito per l'operato faticosamente svolto. Colleghi senatori, sappiamo tutti che la situazione di crisi e gli obiettivi di crescita del nostro Paese ci impongono, tra le tante necessità, quella di rinnovare il sistema scolastico in modo tale da renderlo più efficiente, e di colmare il baratro esistente tra la scuola e il mondo del lavoro. Per la prima volta dopo decenni si sta seriamente lavorando in questa direzione, per il bene dei nostri figli e del nostro Paese. Non lasciamo - è questo il mio invito - che le divisioni e le critiche preconcette ostacolino tale percorso. Andiamo avanti sulla strada intrapresa. Lavoriamo insieme per restituire alla scuola italiana lo standard che essa merita. sull'informativa del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, onorevole Gelmini, che ringrazio, a nome dell'Assemblea, per la disponibilità dimostrata. Onorevoli colleghi, previ accordi intercorsi tra i Gruppi, gli interventi sull'episodio di violenza che ha riguardato una famiglia di origine pakistana in Provincia di Modena si svolgeranno domani mattina in apertura di seduta. Seguiranno gli interventi su alcune dichiarazioni pronunciate dal senatore Ciarrapico giovedì scorso, in occasione del dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio. In entrambi i casi, i Gruppi avranno a disposizione cinque minuti ciascuno. Si passerà poi all'esame dei disegni di legge in materia di divieto di propaganda elettorale e di potestà genitoriale.

il diritto di intervenire, perché si riapre il dibattito. Questo è un fatto regolamentare e, quindi, è solo questo il problema.

non siamo in sede di esame di un disegno di legge. Io non ho la pretesa di conoscere il Regolamento dell'Aula come lei, faccio solo presente che il Ministro ha ascoltato una serie di interventi, ed io la ringrazio di questa attenzione prestata verso tutti. Da parte mia vi è l'impegno a non intervenire, ma non posso parlare per tutti perché mi arrogherei un ruolo che non mi appartiene.

nostra organizzazione dei lavori e su come stanno andando le cose: senza vincolo di mandato, come senatore semplice, perché decidono i Capigruppo. Ciò non di meno,

Noi lavoriamo molto intensamente sui decreti del Governo e, forse, potremmo programmare i nostri lavori in modo tale che quel grande lavoro ispettivo (perché ognuno di noi è depositario di tantissime interrogazioni, anche in Aula) trovi modo di esplicitarsi. Se continua questo susseguirsi di pause vuote e di non intensissimi lavori d'Aula, noi potremmo programmare con il Governo - anche se so che non è facilissimo - una - una risposta sollecita, attenta e rispettosa alle montagne di interrogazioni che tutti i senatori hanno, di volta in volta, depositato. Insomma, so che vi sono i Regolamenti da rivedere e così via, ma dovremmo organizzare un

Signor Presidente, è notizia di oggi che un giovane uomo di 38 anni, laureato in economia e commercio, dopo innumerevoli tentativi di trovare un'occupazione e dopo l'ennesimo viaggio della speranza dal suo paese d'origine, Ostuni, in Puglia, fino a Milano, non riuscendo più a sostenere la situazione si è lanciato da un treno in corsa. Purtroppo, non è il primo caso di suicidio per assenza di lavoro di cui abbiamo notizia in questi ultimi tempi. È sempre notizia di questi giorni che, finalmente, dopo ben 153 giorni di *interim*, il Presidente del Consiglio ha nominato il nuovo Ministro dello sviluppo economico. Senza nascondere il disappunto per l'ennesimo conflitto d'interessi che questa nomina comporta, chiedo al ministro Romani di lavorare da subito ai numerosi *dossier* di aziende in crisi che da mesi giacciono inevasi presso il suo Dicastero e di mettere immediatamente in cantiere, di concerto con il ministro del lavoro Sacconi, politiche davvero concrete per arginare l'altissimo tasso di disoccupazione in Italia. Questa crisi sta mettendo a dura prova gli italiani, e la mancanza di prospettive future per tanti giovani si sta traducendo, purtroppo, in gesti eclatanti sempre più autolesionistici. Il Governo non può più rimanere insensibile davanti a queste tragiche richieste d'aiuto, destinate a moltiplicarsi a causa del protrarsi della crisi e dell'assenza, fino ad oggi, di risposte adeguate. Per questo, signor Presidente, chiedo un intervento da parte dei due Ministri. Senatrice Carlino, la Presidenza prende atto della sua richiesta.